l'A.S. 1880-A, a dispetto del titolo che fa riferimento a «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»,

stesso. Nella mattinata di oggi, dopo il rinvio da lei disposto e deciso in Conferenza dei Capigruppo *ex* articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato, la Commissione giustizia si è riunita per l'esame del provvedimento sul cosiddetto processo breve. In quella sede, pur essendosi sviluppata una discussione nel corso della quale le opposizioni chiedevano che venissero esaminati e votati i subemendamenti presentati dai componenti dell'opposizione, la decisione della Presidenza della Commissione è stata di non procedere a tale esame Questa situazione, questa evenienza, non è nuova nella storia del Senato. In una nostra ricerca, sia pure ancora frettolosa, abbiamo trovato due precedenti analoghi. Ci troviamo cioè di fronte a due identici casi nei quali la Commissione torna ad occuparsi di un provvedimento *sub specie* di emendamenti che sono stati presentati direttamente in Aula, sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, su disposizione del Presidente del Senato. Nel primo caso,

Pastore), si avvia una discussione tra i componenti della maggioranza e i componenti dell'opposizione e, alla fine, si decide di procedere alla votazione dei subemendamenti agli emendamenti che sono stati presentati L'altra vicenda è ancora più interessante sotto il profilo dell'interpretazione del Regolamento e della prassi parlamentare. Ci troviamo di fronte ad una discussione che riguarda un decreto-legge; il Ministro competente è il ministro Maroni. Vengono presentati in Aula degli emendamenti del Governo e lo stesso ministro Maroni richiede, per un approfondimento ed una valutazione di questi emendamenti, il rinvio del provvedimento in Commissione. Il Presidente di turno dispone il rinvio del provvedimento in Commissione, ai sensi dell'articolo comma 11, del Regolamento, e, anche in quella sede, si procede ad una votazione. Mi sembra quindi che la decisione di oggi si ponga - almeno rispetto a questi precedenti, ma è possibile che, se la ricerca fosse stata più accurata, ne avremmo trovati degli altri - in contrasto con una prassi precedente del Senato. La questione è di particolare importanza (voglio ribadirlo in questa sede, anche rispetto ad un argomento che ho adoperato nella giornata di ieri), perché essa riguarda la prassi di presentazione in Aula di emendamenti

ma anche il Presidente della Repubblica - è che i decreti-legge che entrano nell'Aula parlamentare con un testo vengono poi stravolti nel proprio contenuto con i cosiddetti maxiemendamenti (che poi possono anche venire sottoposti al voto di fiducia), con una evidente, palese e chiarissima espropriazione nei confronti dell'opposizione, dell'Aula e del Senato nelle sue diverse articolazioni della possibilità di valutare, emendare ed approvare il testo avendone avuto una piena conoscenza. Questa è la ragione per la quale, signor Presidente, con riguardo a ciò che è avvenuto oggi in Commissione giustizia, le chiedo di convocare la Giunta per il Regolamento per decidere definitivamente sulle procedure da seguire in Commissione, dopo il rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, con riguardo sia ai disegni di legge che ai decreti‑legge, atteso che la prassi di votarne il contenuto è ormai

in Commissione sugli emendamenti presentati e li ha illustrati, sottolineando come gli emendamenti fossero il portato di indicazioni venute dalla Commissione nel corso della discussione che si era tenuta nei giorni precedenti. Successivamente i colleghi dell'opposizione hanno rappresentato l'opportunità che si considerasse quella rimessione alla Commissione come una fase referente e di conseguenza venissero valutati e votati i subemendamenti presentati. Nel solco dell'indicazione puntuale e precisa che la Presidenza aveva fornito,

dell'atteggiamento da adottare è stato letto il documento che lei, signor Presidente, aveva redatto, il provvedimento che lei aveva emesso. Poi il Presidente della Commissione ci ha comunicato l'interpretazione autentica del documento medesimo, dopo aver comunicato con lei,

è stato contrario alla loro proposta di discutere, esaminare e votare i subemendamenti e, con un atto che ci ha profondamente turbato sul piano personale e professionale, perché avremmo gradito vivamente

Si è presa in considerazione tutta la situazione e alla fine il Presidente ha sconvocato la

della decisione dell'opposizione, perché sono certo che, nel corso del dibattito che ci sarebbe stato, ulteriori argomenti utili a una più proficua e virtuosa elaborazione del testo legislativo in esame. Tra l'altro, desidero sottolineare in questa sede, avendone l'opportunità, che nella stesura degli emendamenti mi sono attenuto

Signor Presidente, avevamo interpretato la sua decisione di stamani di rinviare gli emendamenti presentati dal relatore come basata sul presupposto, da lei stesso enunciato, che gli emendamenti del relatore avessero un contenuto

Sulla base di questo, interpretando il nostro Regolamento,

dei poteri tipici di una Commissione e non si trasformasse in un luogo di mera riflessione, dove tra noi, per poi affidare al buon cuore - sicuramente diligente e sensibile - del relatore Valentino la possibilità di interpretare le nostre riflessioni.

Sicuramente le nostre osservazioni e proposte sarebbero state soccombenti nel voto in Commissione, ma sarebbe stato quello l'*iter* corretto;

divergente rispetto alle prassi attuate in precedenza, che ha assegnato alla Commissione un ruolo anomalo, quasi fosse un luogo di riflessione, una sorta di pensatoio, senza che lo stesso potesse approdare a nulla. Abbiamo molto apprezzato la sua decisione di investire la Commissione, attesa la delicatezza della materia;

nei suoi lavori soltanto perché venti persone devono riunirsi per parlarsi su un emendamento senza dover prendere posizione su di esso in modo formale?

poi distorta nell'applicazione di quell'invito che lei aveva fatto alla Commissione giustizia del Senato. se dovessero residuare dubbi interpretativi di una visione dinamica e anche concreta

su un'interpretazione del Regolamento che tenga conto delle prassi abbastanza recenti sia comunque una strada che assegna a tutti quanti la tranquillità di aver fatto un buon lavoro nell'interesse dell'istituzione che rappresentiamo e non esclusivamente un passaggio inutile

perché è chiaro che la decisione che lei ha assunto oggi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 non poteva e non doveva essere più ampia di quello che è stato considerato che è una decisione che ha assunto nella sua qualità di Presidente del Senato,

Devo dire per la verità, al di là della questione del precedente di cui parlerò, che probabilmente se ieri si fosse acceduto alla tesi di un rinvio in Commissione del provvedimento noi avremmo perso meno tempo e stasera ci saremmo ritrovati esattamente qui, a quest'ora, ad iniziare l'esame puntuale del disegno di legge senza sprecare tutto questo tempo, che sarebbe stato forse più utilmente impiegato. Ora, signor Presidente, il problema è la sua decisione, che mi rendo conto è servita in qualche modo ad agevolare il dibattito, il confronto aspro tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, non poteva però che essere viziata all'origine dai limiti entro cui poteva essere adottata, perché in realtà si è trattato di fatto di un rinvio del provvedimento in Commissione, considerato che gli articoli cui fanno riferimento gli emendamenti del relatore sono tre su

formalmente all'esame della Commissione solo ed esclusivamente - almeno così abbiamo letto e discusso in Commissione - gli emendamenti del relatore, è chiaro che ciò si è prestato e si poteva prestare a più interpretazioni,

lasciamo stare se con il voto o meno degli emendamenti - ma senza la possibilità di avere un mandato pieno di esame, di approfondimento di tutte le questioni che riguardano gli articoli interessati dagli emendamenti del relatore. Quando parlo di tutte le questioni mi riferisco a quelle introdotte a seguito dell'emendamento del relatore, con riferimento non solo ai subemendamenti che sono stati presentati prevalentemente, se non esclusivamente, dai Gruppi di opposizione, ma anche con riferimento agli emendamenti che su quegli articoli i Gruppi hanno presentato e che ovviamente trattano anche questioni che non sono state dedotte nella discussione in Commissione dagli emendamenti del relatore. Quindi, al di là della questione relativa al voto o non voto sugli emendamenti e al precedente che è stato richiamato, l'approfondimento e la discussione avrebbero dovuto comunque riguardare la totalità delle questioni sollevate con il maxiemendamento del relatore, non fosse altro che per venire incontro all'esigenza - questa sì limitata e formale

Presidente, in Commissione giustizia c'è stata una vivace discussione

Le debbo dire, signor Presidente, che da parte della maggioranza e del Presidente della Commissione

ai colleghi dell'opposizione, né a quelli della maggioranza, di entrare nel merito degli articoli, e magari di illustrare surrettiziamente i subemendamenti, alla luce dell'illustrazione da parte del senatore Valentino dei nuovi emendamenti Questo è tanto vero che, dopo la decisione legittima dei colleghi dell'opposizione di abbandonare i lavori della Commissione, si è proceduto all'illustrazione - in alcuni passaggi anche critica degli emendamenti presentati dal relatore. Ci siamo trovati dunque nella necessità di esaminare gli emendamenti del relatore,

il mandato ad esaminare soltanto ed esclusivamente gli emendamenti del relatore: non si parla né degli altri emendamenti presentati dai senatori, nè dei subemendamenti. Il motivo per cui è stata decisa la trasmissione degli atti alla Commissione è stato proprio quello di consentire al relatore - che non aveva potuto farlo in Aula - di illustrare i propri emendamenti presentati, appunto, per l'Aula.

seguendo la richiesta che mi era stata fatta dal collega Legnini, mi sono permesso di interloquire con lei per avere da lei una sorta di interpretazione autentica di quello che sembrava peraltro facilmente interpretabile. Alla luce di quanto sopra, abbiamo sottoposto La maggioranza ha ritenuto di respingere quella proposta; si è proceduto quindi all'illustrazione, come ha ricordato il senatore Valentino, del relatore ed anche allo svolgimento di critiche costruttive per rendere quel testo migliore. Abbiamo quindi ottenuto - non dalla benevolenza del relatore, ma dal dibattito che c'è stato in Commissione accoglimento sostanziale di alcune proposte emendative che ci siamo permessi di presentare. Se i senatori dell'opposizione fossero rimasti in Commissione, certamente saremmo stati in grado di svolgere proficuamente quel lavoro che ci era stato consegnato: avremmo potuto illustrare, criticare e proporre modifiche a quegli emendamenti facendo quindi un servizio all'Aula di Palazzo Madama.

Questa mattina, nell'ottica di condurre questo dibattito ad un clima più pacato, questa Presidenza si è assunta la responsabilità di applicare 100 del Regolamento. Era una responsabilità esclusiva della Presidenza - così recita il Regolamento - di trasmettere gli emendamenti del relatore alla Commissione. Sull'*iter* che deve seguire questa scelta vi sono, mi riferisco alla senatrice Finocchiaro e ad altri colleghi, percorsi diversi che vanno in sensi opposti. In alcuni casi, la Commissione ha deciso di muoversi in sede referente, in altri si ha proceduto ad un approfondimento del dibattito. Voglio dire che non vi è un consolidato, né in un senso, né nell'altro. In questa occasione la Commissione ha deciso con un proprio voto, assumendosi quindi la responsabilità della scelta di percorso, di non procedere alla fase referente bensì ad un approfondimento di emendamenti che erano stati trasmessi ad essa da parte della Presidenza.

l'interpretazione può prestarsi a varie ipotesi, e proprio per questo mi riservo, non certo in questo momento, di richiedere alla Giunta per il Regolamento un'interpretazione, sapendo che in questo momento il deliberato della Commissione giustizia si è posto su una prassi di altri precedenti: possono essere condivisibili o meno, ma vi sono state analoghe interpretazioni e scelte. Quindi, inviterei inviterei i colleghi ad andare avanti nei lavori, perché è giunto il momento di continuare nell'illustrazione delle pregiudiziali. Mi spiace che il mio invito ad approfondire in Commissione dei temi delicati

Presidente, molto opportunamente lei richiama il deliberato all'unanimità della Conferenza dei Capigruppo ed io sono qui a confermarle la lealtà del Partito Democratico rispetto a quel deliberato. Voglio però ricordarle che la lealtà è un sentimento - se così posso chiamarlo - bilaterale,

e ricorderà come, da parte di tutte le opposizioni, siano state messe in rilievo, in modo puntuale, le ragioni costituzionali, regolamentari e anche politiche che hanno portato le opposizioni a chiedere che il provvedimento tornasse in Commissione, dal momento che era stato innovato praticamente nella sua totalità. Lei certamente ricorderà quale fosse lo spirito che sorreggeva questa nostra richiesta.

e sia lui che il presidente Berselli hanno riferito di aver chiamato il Presidente del Senato per chiedere delucidazioni su come comportarsi. Io immagino che il Presidente del Senato abbia dato le delucidazioni che gli sono state richieste

noi abbiamo chiesto ieri, e chiediamo oggi, che vengano rispettati i nostri diritti! Noi non stiamo chiedendole del merito! Del merito, e sul merito, finora non si è detta una parola.

Così stanno le cose. Io non do prescrizioni alla Commissione. Conosco il Regolamento e, se il Regolamento fosse stato vincolante, avrei detto al presidente Berselli che era obbligato a seguire un percorso. Questo, però, non è previsto. ZANDA *(PD)*. Presidente, noi le abbiamo citato dei precedenti e comunque... PRESIDENTE. Anche perché, scusi se la interrompo, siccome avevamo fissato un orario per riprendere i lavori,

Io ho sentito in Aula il relatore e il Presidente della Commissione dire che si sono consultati con il Presidente del Senato. Cosa ha fatto il Presidente del Senato? Come oggi ho sottolineato

Io le chiedo soltanto di rispettare i diritti dell'opposizione!

Signor Presidente, credo che a questo punto sia giusto raccontare la storia del confronto che c'è stato tra la maggioranza e l'opposizione sulla calendarizzazione di questo provvedimento. Io capisco la necessità dell'opposizione di farsi sentire e di cercare la massima visibilità per mostrare la propria azione di contrasto a questo provvedimento: sono spinti dai giornali, domani hanno bisogno di vedere... domani hanno bisogno di vedere... Io non ho interrotto il senatore Zanda; voi, se volete, interrompetemi pure, ma credo di dover continuare il mio intervento. Avete bisogno della vostra visibilità, perché è chiaro che state portando avanti un'azione politica

colleghi. BRICOLO *(LNP)*. Voglio semplicemente rendere partecipe l'Aula del confronto che c'è stato fra maggioranza e opposizione sulla calendarizzazione di questo provvedimento. Allora, credo che sia giusta comunque la volontà di farsi sentire e la ricerca di visibilità; ieri sera abbiamo visto come vi siete posti nei confronti dell'Aula, diciamo in maniera poco ortodossa. *(Commenti

adesso elencherò, Presidente. Potevamo, come maggioranza, chiedere la calendarizzazione di questo provvedimento nel mese di dicembre, e non l'abbiamo fatto. Abbiamo, in due occasioni, raddoppiato i tempi di discussione per le opposizioni perché era stato chiesto in Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo posticipato di una settimana la votazione finale di questo provvedimento per permettere alle opposizioni di esprimersi al meglio in quest'Aula. Abbiamo ceduto i nostri tempi alle opposizioni, come richiesto, per dare loro più tempo di discussione; tempo di discussione; abbiamo allungato i termini di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore, perché non li avevate presentati nella giornata di ieri; abbiamo fatto, evidentemente, una serie di concessioni che, a mio modo di vedere, non giustificano e rendono inammissibile l'ostruzionismo in Aula di fronte alla disponibilità da parte della maggioranza a confrontarsi

Presidente, vorrei soltanto, con pacatezza, reagire a una ricostruzione dei fatti che non convince e, soprattutto, che può essere verificata da tutti coloro sono stati interpreti di questi momenti.

sollecitazioni affinché potesse esservi un approfondimento dei temi e un approfondimento delle questioni. È stata una decisione assunta tenendo conto della rilevanza delle tematiche e delle sollecitazioni che sono provenute dall'opposizione. Nella giornata di ieri è accaduto che

Signor Presidente, non sarò io, che sono molto meno parlamentarista dei miei colleghi dell'opposizione, che ritengo che tra Governo e maggioranza ci sia una solidarietà,

e che il Parlamento avrebbe dovuto attendere quella decisione, come lei giustamente ha fatto notare all'Assemblea. Da parte nostra, infatti, ci possono essere anche delle inclinazioni istituzionali che vanno più in un senso o nell'altro, ma questo non è consentito al Presidente del Senato che deve invece garantire la centralità del Parlamento, almeno fino a quando questa Carta e questi Regolamenti lo governeranno.

il Capogruppo della maggioranza l'ha richiesta laddove era stata negata, ma perché nel momento nel quale anche il Capogruppo della maggioranza l'ha richiesta c'era un'unanimità: c'era una richiesta che veniva sia dall'opposizione che dalla maggioranza.

di questo Parlamento e del Presidente del Senato che, anche in questo caso, non ha fatto nessuna preferenza; ha semplicemente seguito una prassi consolidata.

forse quanto sta accadendo in quest'Aula può spiegarsi alla luce di ciò che lei ci ha detto ieri sera, verso il termine della seduta. Leggo dal resoconto stenografico: «La polemica politica (...) la si faccia altrove, non in quest'Aula». Ora, poiché non possiamo credere che lei abbia inteso rievocare il motto di infausta memoria «qui si lavora, non si fa politica», le chiediamo: che cosa stiamo a fare qui?

La Presidenza, *pro bono pacis*, proprio per garantire i diritti dell'opposizione e non dare la sensazione che fosse preclusa tale richiesta, ha esaminato il Regolamento, ha visto che vi era l'ipotesi di trasmissione, non del disegno di legge, ma di singoli emendamenti (quelli del relatore), ed ha concordato,

concluso per mercoledì alle ore 12, perché c'è una richiesta di diretta televisiva). Tutto questo avveniva in un approccio abbastanza responsabile da parte di tutti, con la mediazione di questa Presidenza, che si è assunta la responsabilità, applicando il Regolamento, di rinviare il provvedimento, per alcune sue parti, in Commissione. È insorta in Aula, adesso, una diatriba sulla interpretazione della norma che si è data la Commissione sull'*iter* dei lavori. Ho chiarito che, quando sono stato interpellato, ho ribadito il concetto che non vi è una prassi consolidata. Colleghi, credetemi, è così: non vi è una prassi consolidata. Se vi fosse una prassi consolidata, io io stesso, così come stamattina ho rinviato il provvedimento in Commissione, direi oggi a voi: vi era una prassi consolidata, è stata violata, ma così non è. Ho ribadito che le Commissioni, in passato, investite ai sensi del comma 11 dell'articolo 100

il comune sentire del fatto che l'Aula venisse investita del voto: l'Aula, che è l'espressione della sacralità del Parlamento, più che la Commissione. La trasmissione degli emendamenti alla Commissione era un gesto di disponibilità della Presidenza, proprio per rispetto per rispetto dei diritti dell'opposizione. Opposizione che questa Presidenza intende quotidianamente rispettare, nonostante eventuali critiche ed eventuali censure, che sono il sale della democrazia, dalle quali non mi faccio intimorire, né in un senso né nell'altro. Non mi faccio condizionare, perché sono in pace con la mia coscienza e ritengo, fino ad oggi, di aver gestito con il rinvio in Commissione, spero saggiamente - posso anche aver sbagliato, sono pronto alle critiche, non mi sottraggo - questa vicenda. A questo punto, però,

decidere il percorso, o se la Commissione, investita dei singoli emendamenti, debba muoversi in sede referente e quindi giungere al voto. Non dimenticando che, poiché l'articolo che ho applicato prevede un ritorno in Aula *ad

rivolgo a tutti, maggioranza e opposizione - se dico che ritengo di aver oggi compiuto il massimo degli sforzi per fare in modo che non si lasciasse un *vulnus* nella storia di questo Senato in questa legislatura, e cioè che una richiesta dell'opposizione di ritorno in Commissione potesse essere resa vana. E ho detto anche in Conferenza dei Capigruppo che applicavo questo articolo assumendomene la piena responsabilità

dalla sensibilità del tema trattato. Il senatore Zanda ricorderà perfettamente che ho motivato il ritorno in Commissione tenendo conto del fatto che si parla di garanzie e di diritti, quindi di un tema sensibile. Quindi, proprio in relazione alla specificità del tema, ho ritenuto di assumermi la responsabilità di rinviare in Commissione questi emendamenti, perché ho motivato nel merito. Poi, onorevoli colleghi, mi appello anche al vostro senso di responsabilità. ha adottato una scelta rispetto ad un'altra in assenza di un Regolamento fisso e perentorio, questo è da approfondire nel prosieguo con un chiarimento e una pronuncia della Giunta per il Regolamento, che possiamo riunire anche la prossima settimana. però, si trasforma questo argomento in acceso dibattito, in contestazioni, in clima esasperato, me ne dorrei moltissimo perché mi renderei conto che evidentemente i miei sforzi, il mio tentativo di ricondurre questo dibattito ad un clima

Capigruppo di maggioranza ed opposizione per consentire all'Aula di continuare i propri lavori sapendo che l'argomento della funzionalità della Commissione, che si vede attribuita

Ha chiesto di intervenire la senatrice Bugnano per illustrare la questione pregiudiziale QP4.

stabiliti nella Conferenza dei Capigruppo. Ora, né la presidente Finocchiaro né il presidente Zanda hanno chiesto di mettere in discussione quella tempistica. Non hanno chiesto di riunire la Giunta per il Regolamento per poi articolare Noi riteniamo che, stante l'estrema importanza del problema che le è stato sottoposto,

la fase successiva si svolge - lei certamente me lo insegna, signor Presidente - o in sede referente o in sede consultiva; poiché la sede consultiva non c'entra nulla con l'esame di merito del provvedimento, si doveva svolgere in sede referente. Se questo non avviene, si viola palesemente l'articolo 72 della Costituzione. Altro che agenzie di stampa! Noi avevamo chiesto ieri, all'inizio della seduta in Commissione per ragioni sostanziali, non perché il Governo si apprestava ad emanare un decreto-legge. E certo non l'abbiamo comunicato noi che si apprestava ad emanare un decreto-legge.

eravamo in presenza addirittura di emendamenti di iniziativa parlamentare, cioè di un emendamento a sua firma, signor Presidente, l'emendamento Schifani (chiamato

esattamente identica a quella che si è svolta in Commissione giustizia questa mattina e a quella che si sta svolgendo oggi pomeriggio in Aula, e la conclusione di quelle Commissioni fu quella che è stata richiamata: può sopprimere il diritto‑dovere di una Commissione di merito di esprimersi con un voto sugli emendamenti e sui subemendamenti. Lei si renderà conto, signor Presidente, della gravità della decisione che ha assunto che ha assunto e che mi auguro voglia rivedere. Tanto più che noi siamo disponibili anche a lavorare giovedì pomeriggio, venerdì e lunedì, se sarà necessario: tutto il tempo necessario per poter votare gli emendamenti e i subemendamenti in Commissione e per poterli poi votare Aula, come prevedono la Costituzione e il nostro Regolamento. Senatore Legnini, ribadisco di aver detto al presidente Berselli che era la Commissione a dover decidere, in assenza di una espressione esplicita del Regolamento; questo mi sono limitato a fare. fare. Confermo il fatto che occorre un approfondimento sull'interpretazione della norma. Proprio per questo ritengo che la mia decisione di proseguire nell'ordine dei lavori non costituisca una violazione del Regolamento: se il Regolamento fosse esplicito e chiaro, mi guarderei bene dal violarlo; non ritengo di aver posto in essere, fino ad oggi, atteggiamenti palesemente offensivi nei confronti di questo Regolamento, che è poi il nostro viatico.

occorre un approfondimento su quello che deve essere l'atteggiamento della Commissione. rispondere alla mia coscienza, per evitare che rimanesse un *vulnus*. Senatore Legnini, le potrei citare centinaia e centinaia di emendamenti interamente sostitutivi, anche di finanziarie, presentati da Governi di qualunque coalizione

faremo a sanare il *vulnus* che c'è stato in questo caso, visto che la Commissione ha operato in modo diverso. Mi dispiace soprattutto dover rilevare che la sua sensibilità, con tutto il rispetto, va a corrente alternata, perché da una parte lei dice che quelli in esame sono temi sensibili, e per questo motivo ha ritenuto di rinviare il provvedimento in Commissione, ma dall'altra non ritiene di dover appurare, con la sua sensibilità, anche questo aspetto, che credo sia altrettanto rilevante, perché sappiamo tutti benissimo che i lavori che si svolgono in Commissione sono altrettanto importanti di quelli dell'Aula, soprattutto in un caso come questo, in cui il provvedimento è stato totalmente stravolto.

stravolto; quindi è anche un po' ridicolo e superfluo il nostro lavoro di illustrazione delle questioni pregiudiziali. È bene però che si sappia quale era la proposta offensiva, nei confronti della giustizia e dei cittadini, che questa maggioranza voleva proporre al Parlamento.

collegando questo risultato al massimo della pena edittale, che il provvedimento prevedeva in dieci anni.

sono reati assolutamente disomogenei, e non v'è chi non veda l'incoerenza e l'irrazionalità di questa elencazione, che contiene quindi una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che ci vuole ovviamente tutti uguali davanti alla legge. Oltretutto, l'articolo 2, con l'idea di collegare la prescrizione processuale alla pena edittale prevista per un reato, confligge anche con disposizioni che promanano da fonti sovranazionali. Mi riferisco in particolare alla normativa collegata alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la corruzione, ratificata dall'Italia nell'agosto del 2009, nella quale si raccomanda agli Stati aderenti di rafforzare la normativa sostanziale e processuale per meglio prevenire e combattere i fenomeni corruttivi. Nel nostro ordinamento giuridico, invece, prima attraverso la legge Cirielli, che ha ridotto i termini della prescrizione del reato, e adesso, con questa normativa che introduce una prescrizione processuale,

l'elencazione dei reati è stata esclusa dall'emendamento presentato dal relatore, mentre si prevede la possibile applicazione della prescrizione processuale a tutti i reati,

*(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è l'ennesimo tentativo di imporre alla produzione legislativa un marchio autoritario, spingendosi fino a rinnegare la sovranità del Parlamento e ad infliggere ferite mortali alla Costituzione. Tre sono i punti della questione pregiudiziale che espongo: a luglio, com'è già stato ricordato, il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione. Ebbene, la previsione dell'estinzione dello strumento processuale anche per i delitti di corruzione cancella i 71 articoli della Convenzione e viola palesemente gli articoli 10 e 11 della Costituzione. È evidente che l'obiettivo di questo disegno di legge, nella misura in cui esso determina la caduta del ricorso ai riti alternativi, portatori di un effetto deflattivo assai significativo, non può essere la celerità del processo, bensì solo la garanzia di passare indenni il processo stesso, facendolo morire. L'incoerenza e l'irrazionalità che contraddistinguono questo provvedimento marchiano in maniera indelebile il testo di irragionevolezza, rivelandone la reale filosofia di fondo. In tal senso, le modifiche annunciate dal relatore, con particolare riferimento all'introduzione dell'estinzione del processo per danno erariale (compresi i processi in corso) e all'estensione del meccanismo estintivo anche ai processi per reati sopra ai dieci anni, mettendo una pietra tombale sugli accertamenti di responsabilità per gravissime truffe (concussione, reati finanziari, usura, eccetera), negano la funzione stessa del processo,

possano estinguere, ad esempio, alcuni processi in corso sui derivati truffa appioppati dalle banche al Comune di Milano. C'è il rischio - ed è già accaduto che vengano salvaguardati gli interessi dei banchieri, dei faccendieri, dei furbetti del quartierino che hanno truffato un milione di risparmiatori, bruciando 50 miliardi di euro di sudato risparmio. euro di sudato risparmio. Proprio oggi a Milano si sta celebrando il processo contro i furbetti del quartierino, con l'ex governatore della Banca d'Italia Fazio alla sbarra per la tentata scalata di Antonveneta. È già accaduto, signor Presidente, che, mentre le associazioni dei risparmiatori raccoglievano deleghe sulla Bipop/Carire (decine di migliaia di è arrivata nei due filoni del processo, a Brescia e a Milano, la Cirielli, che ha estinto i processi e ha ammazzato il diritto dei risparmiatori ad avere giustizia. Per questa ragione chiediamo che non si passi all'esame del provvedimento

La volontà dei sostenitori di questo provvedimento non è quella di affrontare e risolvere una problematica allarmante per il Paese, bensì quella di contestare e contrastare le decisioni del potere giudiziario, tirando in campo le tanto disattese raccomandazioni della Corte di Strasburgo e le innumerevoli condanne da essa inflitte all'Italia, al solo fine di giustificare un semplice, quanto subdolo, strumento *ad personam*. La dimostrazione lampante di un tale intento sta nella strana dimenticanza, da parte del Governo, della maggiore flessibilità già accordata nel disegno di legge n. 1440, in corso di esame in Commissione giustizia del Senato, alla durata del processo di primo grado, nella misura in cui esso ritiene come non irragionevole una durata non eccedente i tre anni. La stessa Corte europea, relativamente alle modalità di indennizzo, ha più volte ribadito l'impossibilità di predeterminare la durata ragionevole del processo, rimandando, alla luce della complessità del procedimento, ad una valutazione caso per caso. Non vi è nel disegno di legge in esame traccia alcuna

Per queste ragioni, tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale QP6, chiediamo all'Assemblea di fermare l'*iter* del disegno di legge n. 1880. Nonostante il Ministro della giustizia dica che l'Europa ci chiede questa riforma, il disegno di legge proposto dalla Commissione viola palesemente la normativa comunitaria e tale violazione rischia di essere aggravata se verranno approvati gli emendamenti del relatore che estendono anche ai reati di mafia e terrorismo il meccanismo di estinzione del processo. La visione che questa maggioranza ha dell'Europa, delle leggi comunitarie e dei nostri obblighi nei confronti

Io non ho dimenticato cosa disse Berlusconi nel suo discorso di insediamento alla Presidenza del Consiglio europeo nel luglio del 2003. Per rispondere a legittime critiche avanzate dal presidente del Gruppo socialista, l'eurodeputato Schulz, lo apostrofò come La risposta di Schulz fu esemplare: «Il mio rispetto per le vittime del fascismo mi impedisce di rispondere». Ecco, oggi, con lo stesso spirito europeista e con la stessa amarezza che colpì l'europarlamentare tedesco, non posso che affermare che, per rispetto delle vittime del fascismo, non metterò sullo stesso piano la legge sul processo breve con le cosiddette leggi leggi fascistissime del 1926. Ma la tentazione - lo ammetto - sarebbe grande. Presidente, il tempo mi impedisce un'illustrazione tecnica, ragion per cui sono costretto a limitarmi ad una nota sintetica. Abbiamo di fronte a noi una manovra a tenaglia che punta all'amnistia permanente: il legittimo impedimento si insegue la prescrizione all'infinito; con il processo breve si cancella il processo Mills, in cui Mills stesso è già stato condannato per essersi fatto corrompere da Berlusconi; con il lodo Alfano costituzionalizzato si cerca il definitivo scioglimento dal vincolo delle leggi, ma il rango costituzionale non impedirà la violazione dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Il partito dell'amore di sé produce una legge *ad libertatem suam* che ghigliottina i diritti di decine di migliaia di parti lese, e persino i processi per strage potranno ad un certo punto essere interrotti dalla chiusura del tempo. Tutto ciò configura l'incostituzionalità del provvedimento in discussione. *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento oggi in esame presenta una serie di problemi generali, senza dubbio gravi. Tre sono le principali criticità del testo oggetto d'esame: la questione dei tempi del processo e, in particolare, la data a partire dalla quale prende il via il computo del decorso temporale; l'applicazione immediata ai processi in corso delle disposizioni contenute nel disegno di legge e, infine, il problema delle sedi di dibattimento. Per quanto riguarda il primo problema, la scelta di fissare a priori la durata di un processo, senza prevedere una valutazione del singolo caso da parte del giudice, contrasta palesemente con la normativa comunitaria. Nel quadro di una siffatta operazione di fissazione e scansione dei tempi del processo, appare contraddittorio il diverso riferimento dei primi due articoli del disegno di legge n. 1880-A alla data di inizio del processo penale, per cui essa coincide prima con la data di assunzione della qualità di imputato, per poi successivamente accogliere anche una fase preliminare al processo *stricto sensu*. Per quanto attiene la questione della retroattività, mi limito solo a segnalare la violazione non solo di un secolare principio in virtù del quale ogni atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui esso si verifica, ma anche dell'articolo 11 delle preleggi. Tale violazione non verrebbe superata, ma, anzi, reiterata ed aggravata se passassero le proposte del relatore, con effetti devastanti anche su processi tecnicamente complessi, come molti di quelli che riguardano il lavoro e la sicurezza dei lavoratori, dei quali ha già parlato la collega Bugnano. È evidente che qui i *vulnus* vanno ben oltre il profilo costituzionale, toccando quello dei princìpi generali. Con riguardo all'organizzazione territoriale dei singoli tribunali, viene in rilievo un problema di discriminazione a carico di quegli imputati che, a causa di ragioni ad essi non imputabili, saranno costretti a vedere scorrere impotenti il decorso del tempo. Nulla è stato previsto per mettere la pubblica amministrazione interessata in condizione di gestire e far funzionare questa "miracolosa" innovazione in maniera imparziale. Per questi motivi e per le ragioni tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale QP8,

e contraddire proprio i principi del giusto processo e della ragionevole durata di cui all'articolo 111 della Costituzione, ai quali dichiara di ispirarsi, nonché la tutela del diritto di azione e di difesa sancito costituzionalmente all'articolo 24. Se il fine è quello di garantire una maggiore efficienza dei procedimenti, non si capisce per quale motivo non sia stata istituita una corsia preferenziale che assicuri maggiore efficienza alla celebrazione dei processi, con particolare riferimento a quelli inerenti i reati di maggiore allarme sociale. Alcun riguardo sotto il profilo della ragionevole durata è riconosciuto, inoltre, alle cause che concretamente incidono sui tempi dei processi; anzi, le modifiche che si prospettano sono tali da aggravare gli effetti già derivanti dall'indulto. dall'indulto. Seguendo la strada indicata dai proponenti e confermata dal relatore, si finirebbe con il fissare termini di estinzione del processo anche per reati riguardanti la sicurezza dello Stato, delitti contro la personalità internazionale dello Stato e reati sui quali abbiamo sottoscritto accordi in sede europea ed internazionale.

finestra") *(IdV)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la discussione che si è accesa negli ultimi giorni sul disegno di legge in esame ha avuto l'effetto di confondere i già poco nitidi contenuti di tale provvedimento. Per i non addetti ai lavori è diventato difficile comprendere quali siano i veri rischi di una tale innovazione nel sistema di giustizia italiano. Il nuovo testo, come ha già rilevato il CSM, introduce una prescrizione processuale che va ad aggiungersi alla prescrizione dei reati, senza tra l'altro prevedere alcuna forma di coordinamento. Nessun Paese dell'Unione europea, signor Presidente, prevede un regime analogo. D'altronde, nessun altro Stato di diritto avrebbe mai deciso di approvare norme così drasticamente lesive dello Stato di diritto. È frutto di un'immaginazione degna dei migliori scrittori di saghe fantascientifiche pensare che in due o tre anni, senza risorse umane e strumentali adeguate, possa svolgersi l'udienza preliminare per poi procedere al dibattimento, all'esame dei testi, comprese le eventuali perizie, e giungere infine a sentenza. Non è bastata la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale a rendere chiaro che la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti; anzi, si prefigura un'ulteriore modifica all'articolo 2 che farebbe rientrare nel meccanismo estintivo anche i reati la cui pena edittale supera i 10 anni, compresi quindi quelli di mafia o magari le stragi. L'articolo 2, già nella attuale formulazione, coinvolge reati-mezzo, solo apparentemente meno gravi, che fanno capo al reato-fine associativo, per i quali la medesima maggioranza auspica anche restrizioni sul fronte delle intercettazioni telefoniche. È lapalissiano, signor Presidente, ribadire che, visto quanto la maggioranza ha già approvato in Commissione e quanto si propone di approvare domani e nei prossimi giorni in questa Aula, l'obiettivo vero non è quello della brevità dei processi. Per queste ragioni,

*(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame introduce un dispositivo mirato a rendere impossibile l'accertamento processuale per intere categorie di reati. Innanzi tutto, sotto il profilo della costituzionalità va rilevato che esso contrasta nettamente con il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione nella misura in cui quest'ultimo dispone che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Il principio della parità delle parti viene totalmente ignorato dal disegno di legge di legge n. 1880-A, in riferimento sia alla questione dell'indennizzo che a quella dell'estinzione processuale. I reati ambientali, gli omicidi commessi per colpa professionale e, se passassero alcune delle modifiche proposte dal relatore, anche i reati sopra i dieci anni, verrebbero letteralmente amnistiati e le vittime subirebbero un'ulteriore e definitiva beffa. Dobbiamo spingerci a insinuare che l'effetto tagliola di questo provvedimento sia stato cogitato al fine di salvare determinati soggetti e condannarne altri in virtù di un criterio di favore sconosciuto? Per queste ragioni, tecnicamente esposte nella questione pregiudiziale n. 11, chiediamo che quest'Aula non proceda all'esame del disegno di legge n. 1880,

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ancora una volta attraverso un disegno di legge siamo chiamati a far fronte ad una situazione di emergenza che attanaglia il presidente del Consiglio Berlusconi. Con riguardo al disegno di legge in esame assistiamo ogni giorno ad annunci, dichiarazioni e *spot* pubblicitari. Di processo di riforma però neppure l'ombra. È chiaro, infatti, che il provvedimento in oggetto non può essere in alcun modo qualificato come strumento di riforma del processo penale, in quanto l'effetto da esso scaturente è quello di falciare i processi e non certamente di renderli più efficienti o più brevi. L'impianto normativo di questo disegno dì legge presenta diversi profili di incostituzionalità, violando gli articoli 3, 10, 24, 111 e 112 della Costituzione. Si è tranquillamente fatto a meno, nella predisposizione del testo oggetto d'esame dei principi della giustizia costituzionale (valga per tutti il criterio del ragionevole bilanciamento degli interessi da proteggere), così come ci si è dimenticati dei criteri comunitari in materia di risarcimento del danno derivante da ingiustificata durata del processo, nonché delle precisazioni della Corte di giustizia europea in merito all'indennizzo che, secondo il giudice comunitario, prescinde dall'esito del procedimento, proprio perché i tempi processuali troppo lunghi, individuati nella durata complessiva del processo e non nella fissazione astratta dei termini indifferenziati per ciascun grado di giudizio, costituiscono in sé una violazione della Convenzione europea dei diritti umani. Un nodo rilevante ai fini dei profili di incostituzionalità è altresì quello della non applicabilità dell'istituto ai giudizi pendenti dinanzi alla corte d'appello o in Cassazione nel momento in cui viene previsto che le norme interesseranno in sede di prima applicazione anche i processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge.

che, sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, c'è stata una condivisione nell'obiettivo di scandire per fasi i tempi del processo

Noi siamo stati e siamo perfettamente convinti della necessità di ridurre i tempi dei processi senza attività normative che si presentano con una motivazione del tutto priva di veridicità. Voi avete avuto il coraggio - e io sostengo che ce ne vuole - di scrivere nel frontespizio la norma che avete presentato: «Misure per la tutela del cittadino» - forse volevate dire: del primo cittadino

farlo attraverso una norma di diritto. Questi sono precedenti gravissimi, destabilizzanti. L'articolo 6 della Convenzione europea e l'articolo 111 della Costituzione italiana richiedono tempi brevi per i processi: mai, in queste norme, si fa riferimento alla morte, all'interruzione del processo come assurda sanzione per il suo protrarsi oltre i termini ragionevoli. Lo Stato italiano si è adattato a queste disposizioni e ha previsto un diritto risarcitorio per la irragionevole durata dei processi; per questo motivo vengono pagati milioni di euro all'anno, e ciò non dovrebbe accadere.

un'eventuale responsabilità disciplinare, che ipotizzo soltanto, perché questo, allo stato dell'arte, non sarebbe possibile. Infatti, tutti voi sapete meglio di me che oggi non è umanamente possibile richiedere a qualsiasi tribunale o a qualsiasi magistrato il rispetto di simili termini; almeno, non in maniera così generica e generalizzata. Noi abbiamo dato prova di senno e di maturità presentando una serie di emendamenti che, se fossero stati accolti, avrebbero dato un senso a questo obiettivo, intervenendo sulle cause per le quali i processi in Italia superano una tempistica ragionevole.

a voi interessa soltanto soddisfare le esigenze immediate del Presidente del Consiglio dei ministri. Si poteva fare, io l'ho detto con chiarezza insieme ai miei colleghi in Commissione giustizia: lo possiamo fare, ma in termini di decenza giuridica, di rispetto per i principi del nostro diritto. Eliminiamo insieme - e la via è chiara

asfittica, incapace di offrire il servizio giustizia al cittadino. Voi con questo provvedimento state negando ai cittadini il diritto di ricevere una risposta giudiziaria, cioè state affossando un diritto sacrosanto, fondato su un valore un valore costituzionale, che è quello dell'accertamento della verità. Con questa legge, pur di soddisfare le esigenze di una persona, voi state impedendo ad un numero indefinito e indefinibile di persone di ricevere la risposta giudiziaria, cioè uno dei servizi più essenziali della democrazia moderna:

probabilmente, e questo è molto grave, non vi consentono di essere liberi e indipendenti. Molti di voi - in questo momento mi astengo dal nominarli, ma lo farò in seguito - sanno bene che ciò che sto dicendo è vero, è fondato sul diritto, e lo condividono;

Parlamento: le stiamo svendendo! Queste norme non servono a nulla o, per lo meno, non servono all'obiettivo che voi indicate anche all'inizio della legge, bensì a tutt'altro. Questo tutt'altro può avere un peso politico e si può perseguire insieme, ma non affossando il diritto, non negando ai cittadini italiani di ricevere una risposta. Ecco perché vi chiedo

una discussione che abbiamo affrontato in precedenza. Essendo stata io oggi artefice, in Commissione giustizia, della decisione di allontanarci dalla Commissione stessa, desidero sottolineare che tale

quello costituzionalmente garantito, e quello delle Commissioni parlamentari. Non c'è stata da parte dell'opposizione altra ragione che questa. questa. Ci tengo a sottolinearlo perché non mi pare di aver colto tale aspetto nella discussione odierna da parte della maggioranza, e questo mi fa profondamente dispiacere perché immagino di partecipare a un Parlamento che ha una sua utilità. Detto questo, vista la brevità del tempo a disposizione, passo ad illustrare la questione che mi induce a chiedere il ritorno in Commissione del disegno di legge e che tocca prevalentemente, per quanto mi riguarda, il tema dei reati in materia di corruzione e dei reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di reati che colpiscono particolarmente la società italiana anche sotto il profilo della criminalità economica economica e della criminalità economica di stampo mafioso. Sono compiuti in larga parte da soggetti che

abbiamo un risultato assolutamente negativo in assenza di una riforma del processo in grado di cancellare duplicazioni di garanzia e abusi di processo, in assenza di dotazioni di mezzi e di risorse perché la magistratura possa e debba funzionare, in ragione della pena edittale prevista in astratto per i reati e, a maggior ragione, in un sistema in cui il codice penale è stato emanato prima dell'entrata in vigore della Costituzione e che quindi si fonda su una scala di valori posta alla base delle sanzioni che ha ormai un carattere anacronistico. Questo profilo resta anche rispetto all'emendamento del relatore poiché rimane un criterio di disomogeneità dei reati in termini di offensività degli stessi calcolato sulla base della pena edittale. Noi ci troviamo quindi, in rapporto al delitto di corruzione, in una situazione che porta necessariamente a far confliggere la previsione della prescrizione processuale sia con la necessità di sconfiggere il fenomeno che costituisce un obiettivo economico e sociale e un momento importante di contrasto alla illegalità e alla criminalità organizzata, sia con la previsione di fonti sovrannazionali che noi dobbiamo oggi tenere presenti sia perché ci siamo impegnati con la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione, sia perché ce lo impongono gli articoli 10 e 117 della Costituzione, sia perché non è risolto l'intreccio tra prescrizione sostanziale (quella del reato) e prescrizione processuale. In conclusione, noi veniamo a violare anche gli articoli 79, soprattutto per quanto riguarda la parte della norma transitoria che finisce con risolversi in un'amnistia, e 112 della Costituzione, che impone l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Il tutto avviene in violazione anche dell'articolo 111 (principio di ragionevolezza) e dell'articolo 24 che contiene il principio generale del diritto alla difesa, depotenziando anche i diritti delle parti offese che, in questo caso, sono la pubblica amministrazione e, quindi, lo Stato italiano. Queste sono le ragioni per cui le chiedo

mi accingo a fare questo intervento in spirito di collaborazione, anche perché ho molta stima per il collega Valentino, relatore sul provvedimento, che avrebbe forse dovuto notare una incongruenza costituzionale abbastanza evidente.

della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni o di quelle sulla circolazione stradale, la prescrizione è di dieci anni.

perché si estingua il reato devono passare ancora quasi cinque anni. Qui sorge un contrasto evidente con l'articolo 112 della Costituzione, con cui si stabilisce

Questo mi pare di un'evidenza solare, ed è stato rilevato anche da eminenti costituzionalisti; mi stupisco che non sia stato notato anche da molti giuristi della della maggioranza, alcuni dei quali hanno fatto riferimento a Leopoldo Elia come a un maestro di tali questioni. Credo che sarebbe stato opportuno verificare soprattutto questa possibilità di contrasto con l'articolo 112 della Costituzione.

Signor Presidente, esiste un problema di ragionevole durata del processo penale nel nostro Paese, così come immaginato dal dettato costituzionale all'articolo 111 e tale da determinare per legge la durata del processo? Forse sì, non mi sentirei di escluderlo; credo che se ne possa parlare ed avevamo iniziato a discuterne. Ce lo ricorda anche l'articolo 6 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come lo statuisce l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal nostro Paese, che ci racconta di un diritto al processo «senza giustificato ritardo», sia nei procedimenti penali che in quelli civili. A tal proposito, vorrei che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa è intervenuto su tale problema con la risoluzione interinale n. 42 del 2009, identificando un totale di 2.183 casi risolti contro l'Italia in merito alla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari. dire che la legge Pinto, nata per porre rimedio a tali carenze del nostro sistema giudiziario, abbia costituito una risposta adeguata ed efficace.

che proprio da questa situazione hanno tratto la spinta e la volontà di procedere a riformare la giustizia nel nostro Paese. Così come del resto non ci sfuggono alcuni dati noti, ripresi da molte fonti e da autorevoli organi di stampa. Partendo proprio dalla legge Pinto: 1.266.000 euro nel 2002, quasi 11 milioni di euro nel 2005, circa 25 milioni di euro nel 2008, 34 milioni di euro per una parte del 2009.

questi dati con quelli di altri Paesi vediamo che in Italia nel 2007 i giudizi penali pendenti in primo grado sono 1.200.000, in Germania 287.000, in Spagna 205.000 e in Gran Bretagna 70.000.

giorni, in Francia 331, in Germania 394. Questa è la situazione, e potremmo continuare a lungo. Ma come abbiamo detto nei lunghi e - a mio avviso - non inutili lavori in Commissione e come ribadiamo oggi, così come siamo consapevoli di come stanno le cose, è altrettanto utile domandarsi se sia ragionevole la risposta che il Senato si appresta a dare in questo contesto e a questo contesto. Pur dando peraltro atto - perché è nei fatti - che ci troviamo di fronte ad un provvedimento sostanzialmente diverso, che tiene conto anche di molte delle proposte emendative da noi formulate, non possiamo considerare ragionevole

seppur succinta, citate. La prima è che non basta accordarsi su un termine se non si pongono in essere le condizioni, i modi, le circostanze funzionali al raggiungimento dell'obiettivo, che deve essere congruo con quello che ci si propone di fare e con la macchina organizzativa, in termini di mezzi, uomini e sedi a disposizione. Se nel 2003 i cancellieri e gli impiegati erano 45.000 e oggi sono 42.000, si può immaginare che ci troviamo invece di fronte alla necessità di colmare vuoti organizzativi e riprendere quindi un discorso di funzionalità della macchina giudiziaria. Del resto, mi pareva che il disegno di legge del Governo presentato nel marzo 2009, e di cui era già stata avviata la discussione generale, fosse la sede più idonea per definire in modo organico la riforma della giustizia e che tenesse quindi conto

in quella norma transitoria in cui il legislatore pare più preoccupato a sanare il passato che non a delineare i confini di un possibile processo penale

per effetto degli emendamenti il suo testo è mutato ma l'impianto e la filosofia del disegno di legge sono gli stessi. Quindi - consentano i proponenti l'ironia - sarebbe meglio espressa questa filosofia cambiando il titolo del disegno di legge. Suggerirei: «Provvedimenti per l'introduzione nella giustizia penale di istituti di diseconomia processuale». Nell'ordito delle nostre norme costituzionali sulla giurisdizione rintracciamo un equilibrio delicato tra la pretesa punitiva dello Stato, la presunzione di innocenza, il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi interessi legittimi del cittadino, ma senza processo o con un processo a conclusione quasi impossibile e sicuramente incerta questo equilibrio non c'è più. articoli 24 e 112 della Costituzione, quest'ultimo relativo all'azione penale obbligatoria, consegnano a noi, al legislatore, il dovere di approntare un sistema che provi a realizzare una nostra umana ed imperfetta giustizia, però un sistema che funzioni, che ragionevolmente possa funzionare, data la sua organizzazione e i mezzi che la Repubblica decide di dedicarvi. Ma se la regola, i mezzi, i tempi del processo rendono oggettivamente improbabile raggiungere lo scopo dell'accertamento della verità - certo, di una verità umana, processuale - questo diritto fondamentale del cittadino, il diritto civile alla giustizia subisce un non rimediabile degrado; e si va contro Costituzione se il diritto alla giustizia, che qui è eminentemente il diritto della parte offesa, il diritto del più debole che può farsi forte solo della forza dello Stato, viene collocato nella zona grigia della non effettività, che è la malattia mortale dei diritti fondamentali. Ecco, senatori, se dichiarassimo solennemente, come dichiara questo disegno di legge, la non effettività del diritto alla giustizia, autorizzeremmo il diffondersi di una grande frustrazione nella catena della giustizia. Come reagirà il primo anello di questa catena, l'apparato dello Stato preposto alla prima cura della legalità, alla dissuasione del comportamento illegale, alla repressione immediata del crimine? Abbiamo chiesto al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, agli avvocati una loro previsione degli effetti. Ma il Ministro dell'interno non ha da dire la sua previsione? Non ci vuole molto ad immaginare l'attività quotidiana delle forze dell'ordine infiltrata dalla grande frustrazione. Molto del loro lavoro, lo sappiamo, sarà reso inutile. sarà compiuto con la stessa diligenza o sarà invece connotato dallo scetticismo, da minore impegno e passione? La *notitia criminis* sarà segnalata, la denuncia del cittadino considerata e con un seguito investigativo o colpirà il pesante messaggio di dissuasione trasportato dal provvedimento in esame? Processo breve incerto, indagini inutili, soldi e fatica sprecati. In conclusione, dissipazione del lavoro di indagine delle forze dell'ordine, dei magistrati, del pubblico ministero, della difesa, delle parti civili e del loro diritto ad un risarcimento diverso da quello monetario. Ecco cosa reca in danno, senza altre misure per la giustizia, il cosiddetto processo breve. «*Fiat iustitia et pereat mundus*», vale a dire «sia fatta giustizia, vada pure in rovina il mondo». Questo era il motto di Ferdinando d'Asburgo. Colleghi, signori della maggioranza, che un giorno non vi si attribuisca a motto della legge che oggi pretendete di imporre al Paese: «Sia fatto il processo breve, rovini pure la giustizia».

Presidente, il modo in cui sono stati organizzati i lavori d'Aula e di Commissione

ad esprimere una serie di considerazioni in ordine alla asserita incostituzionalità di un testo che, nottetempo, è stato radicalmente modificato e che verosimilmente sarà approvato nella stesura proposta dal relatore e non nella nella stesura licenziata dalla Commissione. È evidente che questo fatto impone dei limiti all'esame dell'Aula. Il primo limite è proprio quello di non consentire all'Assemblea di esprimersi compiutamente sui profili di incostituzionalità

testo, frutto della scelta della maggioranza di non consentire un corretto esame istruttorio del provvedimento in Commissione. Si tratta di un profilo di incostituzionalità per un vizio del procedimento legislativo, che peraltro reiteratamente il Capo dello Stato in più occasioni (da ultimo, con riferimento al cosiddetto pacchetto sicurezza) ha avuto modo di sottolineare, in maniera estremamente rispettosa dell'autonomia e delle prerogative del Parlamento, sintetizzandolo nella necessità della trasparenza dell'azione del legislatore, dell'intelligibilità dei testi normativi e della loro accessibilità da parte di chiunque, di ogni singolo cittadino, indipendentemente dal fatto che si tratti di un addetto ai lavori o meno. A questo punto, non riesco neanche a capire cosa ci stia fare nel Governo un Ministro per la semplificazione, se poi siamo costretti a votare norme di questa questa natura, che non hanno alcuna accessibilità e comprensibilità e che sono state costruite appositamente in questo modo per nascondere le ragioni per le quali sono state proposte ed approvate. Limiterò pertanto le mie osservazioni, signor Presidente, a quelle parti del testo che resistono al maxiemendamento del relatore e, e, per economia dei nostri lavori, svolgerò alcune considerazioni sui profili di incostituzionalità, che, dal nostro punto di vista, anche il testo proposto dal relatore ha e porterà con sé nel suo successivo *iter* parlamentare.

della cosiddetta ragionevole durata dei processi civili, amministrativi, eccetera, ai fini della costruzione della condizione per l'esercizio dell'azione relativa al diritto all'equo indennizzo, sono quelli del testo della Commissione. Si tratta di termini ridotti

a fronte di 5.425.000 processi civili, il 50 per cento di essi sarà colpito da queste norme. Per quanto riguarda i giudizi amministrativi, quelli pendenti da più di due anni sono 566.339 in primo grado e oltre 23.000 in secondo grado, considerando le sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda i giudizi davanti alla Corte dei conti, quelli colpiti sono circa 38.000. Poiché con queste norme che introducete il decorso del termine costituisce causa unica*, ope legis*, per la richiesta del diritto all'equo indennizzo, è evidente che la sovraesposizione finanziaria del bilancio del Ministero della giustizia è tale che necessita di una quantificazione e di una copertura, ai sensi dell' articolo 81 della Carta costituzionale. Non vi siete però limitati a questo, perché nell'emendamento proposto dal relatore avete introdotto un doppio grado di giudizio, sotto forma di opposizione al decreto presidenziale, e quindi un riesame dell'eventuale decreto motivato del presidente o del consigliere delegato che respinge o accoglie la domanda di equo indennizzo, che di fatto, che di fatto, a fronte della mole di contenzioso che si svilupperà sull'applicazione della legge Pinto, appesantirà così tanto i giudizi pendenti davanti alla Corte d'appello da rendere oggettivamente impossibile celebrare in tempi ragionevoli i giudizi sull'equo indennizzo. Questo è il paradosso al

Su tale aspetto avete sostenuto e continuate a sostenere, con una bella faccia tosta, che comunque tale tutela è garantita anche a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio, perché c'è la possibilità della trasposizione in sede civile dell'azione, che la parte civile ha già a prescindere, e che tutto questo avverrebbe con una rimodulazione delle priorità nel calendario per la celebrazione dei giudizi che le riguardano. Tutto questo sulla carta va benissimo, ma quando passiamo dalla carta cioè dalla realtà che vi siete costruiti, dalla vostra finzione - alla realtà, ci rendiamo conto che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Occorre infatti considerare che lo stato di

più efficiente la celebrazione dei processi civili, con buona pace dei riti alternativi e delle miniriforme che sono state introdotte, che, essendo facoltative, non produrranno gli effetti che sperate o dite di sperare. Tutto questo Tutto questo determina una crescita esponenziale del contenzioso e quindi determina di fatto una previsione normativa illogica e che, anziché perseguire l'obbiettivo che si è posto, ne persegue uno esattamente opposto: quello di rendere ulteriormente irragionevoli questi giudizi. Con riferimento alle vittime di reato, si nega loro la possibilità di avere il ristoro morale ‑ e non solo quello che nasce dall'azione risarcitoria di stampo civile ‑ nella sede propria, che è il processo penale,

la questione dell'azione e dell'introduzione da parte del relatore della prescrizione del processo contabile. Al di là dell'assoluta irragionevolezza

Ditemi voi come si fa a stabilire se un giudizio contabile si estingue in ragione di due o tre anni, a seconda che il pubblico ministero (il procuratore, nell'azione della Corte dei conti) stabilisca che

pubblica. È quindi evidente che il computo dell'attività istruttoria nell'ambito della durata complessiva di un giudizio di due o tre anni determinerà di fatto una compressione dei diritti di difesa del convenuto,

questione, è evidente che il risultato finale di questo papocchio sul giudizio contabile sarà che la Corte dei conti in primo e secondo grado procederà a condannare sullo stato degli atti, senza andare ad accertare la veridicità delle contestazioni, perché non avrà il tempo di farlo. Poiché ciò che prevale è l'interesse statistico alla consumazione di determinati giudizi, alla fine la compressione avverrà sui diritti di difesa, con buona pace di quanto andate dicendo in giro. Da ultimo, signor Presidente,

anzi, questa coda di amnistia sotto forma di indulto, così come l'avete costruita al comma 1 dell'articolo 4-*bis* - è veramente esilarante, e tralascio le ragioni per cui ciò è stato fatto.

L'interpretazione del testo che lei ha proposto comporta la circostanza della durata ultrabiennale che, per i delitti indultabili e per i reati coperti da indulto o che possono essere soggetti ad indulto, riguarda

che sono oggetto di accertamento giudiziario in primo grado e che superano i due anni ma tutti i processi che riguardano quelle ipotesi di reato il cui giudizio di primo grado dura più di due anni. Se fosse così, al di là della incostituzionalità, ci troveremmo di fronte ad una abnormità

per cercare almeno di ottemperare all'invito del Capo dello Stato. Non lo potete fare a chiacchiere e poi dimenticare ciò che in quest'Aula viene detto: della pausa estiva, sul pacchetto sicurezza questa maggioranza, questo Governo e - lo dico senza polemica - la Presidenza del Senato altro hanno detto rispetto alla lettera garbata del Capo dello Stato che ha posto alcune questioni essenziali per il ruolo di questo Parlamento, che voi quotidianamente state mortificando.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato con attenzione le 27 questioni pregiudiziali e sospensive presentate dall'opposizione credo che serva da parte nostra una breve replica, soprattutto con riferimento ad alcuni passaggi contenuti in tali questioni pregiudiziali, che contengono errori anche di carattere tecnico. Si è detto anzitutto che nel nostro ordinamento interno non esisterebbe l'istituto della prescrizione processuale, e quindi che questo meccanismo estintivo sarebbe introdotto per la prima volta; in particolare, la questione pregiudiziale QP9 dell'Italia dei Valori dice espressamente che l'istituto della prescrizione del processo è sconosciuto all'ordinamento interno. Purtroppo non è così e molti di voi lo sanno perché il processo disciplinare nei confronti dei magistrati prevede la prescrizione processuale. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede un termine fisso di due anni per la durata del processo disciplinare affidato alla sezione disciplinare del CSM

che la ragionevole durata del processo disciplinare nei confronti di un magistrato sia di due anni, senza alcun riferimento alla maggiore o minore gravità dell'illecito disciplinare del magistrato stesso. Solo due anni. Per i magistrati il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è stato attuato e all'indeterminatezza del concetto di durata ragionevole del processo si è sostituito un termine definito e certo *ex ante;*

che è l'organo consultivo costituito in seno al Consiglio d'Europa, che si occupa di misurare e di valutare l'efficienza dei vari sistemi giustizia nei diversi Paesi membri - ha approvato Paesi membri - ha approvato un documento, denominato Programma Quadro, dal titolo «Un nuovo obiettivo per i sistemi giudiziali: la trattazione di ciascun caso entro una cornice temporale ottimale e prevedibile». Quindi, il Consiglio d'Europa, con il suo organo consultivo, prevede che «ogni processo deve svolgersi entro un limite temporale non semplicemente ragionevole, bensì ottimale e prevedibile *ex ante*».

Aggiungo poi che il tema della prescrizione processuale e dei meccanismi estintivi nel 2008 era stato addirittura proposto dall'Associazione nazionale magistrati al ministro Alfano, al momento del suo insediamento.

endoprocessuale. In verità, colleghi dell'opposizione, a voler essere sinceri fino in fondo, l'unica critica seria che poteva essere fatta a questo provvedimento è che esso è stato copiato dai disegni di legge del centrosinistra: questa è l'unica critica seria che poteva essere

e che è pertinenza assoluta del mondo dei giuristi di centrosinistra. Se qualcuno avrà la cortesia di leggere un bellissimo libro del 2003 dei professori Giunta e Micheletti sulla prescrizione processuale, si accorgerà che vengono

senatore Fassone, in un articolo su «Questione giustizia» del 2001, a proposito dell'introduzione della prescrizione processuale diceva: «La magistratura non solo non sarà incoraggiata a sonnecchiare, ma sarà sollecitata ad attivarsi sin dalle prime battute, e la durata del processo non sarà indefinita, ma sarà frutto di una somma di addendi ben definiti e serrati tra loro». A noi piacerebbe davvero che in quest'Aula ci fosse ancora il senatore Fassone.

le questioni pregiudiziali che sono state poste sono in buona parte riconducibili ad argomenti che non sono quelli reali. Si chiede, ad esempio, il rinvio in Commissione

disposto l'ulteriore esame in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, per cui questo ulteriore esame c'è stato, e poi ricordo che non siamo in sede redigente, cioè quella sede in cui la Commissione approva l'intero testo e poi l'Aula si limita alla votazione degli articoli ed al voto finale; pertanto è certamente legittimo chiedere di ritornare in Commissione, nel senso di essere contrari all'approvazione del provvedimento, ma l'esame in Commissione c'è stato. Dico di più: gli emendamenti proposti dal senatore Valentino non nascono dal nulla ma dal dal dibattito che si è svolto in Commissione giustizia; aggiungo che accolgono le condizioni e gran parte delle osservazioni prospettate dalla Commissione affari costituzionali quando ha espresso il proprio parere per quanto riguarda le materie di propria competenza su tale provvedimento. Un secondo punto che vorrei sottolineare è il seguente. Da certi interventi sembra la prescrizione sarebbe quasi introdotta da questo provvedimento, come se oggi non ci fossero processi che vanno in prescrizione.

Tant'è vero che questa esigenza è stata sentita nel passato soprattutto da autorevolissimi esponenti del centrosinistra, i quali, come ricordava il senatore Mazzatorta, hanno

molto efficace l'effetto che queste nuove norme dovrebbero avere sui processi in corso. Questo è un aspetto sul quale molti degli interventi dell'opposizione si sono soffermati. Vorrei ricordare in merito che cosa diceva il disegno di legge presentato dai senatori Fassone, Ayala, Brutti, Calvi e Maritati, tutti uomini di diritto di notevole livello. Nella relazione al loro disegno di legge ricordavano che sembra inevitabile pervenire alla conclusione che nei procedimenti in corso il termine di prescrizione sarà quello risultante in concreto più vantaggioso per l'imputato, a seconda che si applichi la disciplina vigente o quella di nuova introduzione, ferma restando l'impossibilità di addirittura contaminare i due istituti nella ricerca di una terza soluzione ancora più benevola dell'una o dell'altra. Per cui non soltanto il contenuto della norma che oggi stiamo esaminando ricalca molto da vicino un disegno di legge presentato da autorevoli esponenti del centrosinistra, in particolare da esperti di diritto (quattro magistrati e un avvocato), ma anche l'impatto di queste nuove norme sui procedimenti in corso è stato chiaramente e succintamente illustrato da queste parole della relazione che ho citato. Credo perciò opportuno proseguire l'esame di tale provvedimento e per questo il Gruppo del Popolo della Libertà voterà contro le questioni sospensive e pregiudiziali.

Colleghi, dobbiamo procedere a tre votazioni: una sulle questioni pregiudiziali, una sulle tre questioni sospensive e una per la richiesta di parere al CNEL.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, è un dato oggettivo e non più un'opinione di alcuni che lo stato della giustizia nel nostro Paese ha raggiunto livelli di inefficienza intollerabili, sconosciuti in altri Paesi democratici, per i quali l'Italia versa da anni in una situazione di illegalità tale da avere generato numerosissime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Corte europea ormai condanna lo Stato italiano per la violazione dei diritti di tutte e di ciascuna parte di un processo: condanne per la violazione dei diritti degli imputati, condanne per la violazione dei diritti delle vittime dei reati e delle parti lese, condanne per la violazione dei diritti dei detenuti. È un fatto che lo Stato italiano non riesce più, e da tempo, a garantire i diritti fondamentali di quei cittadini che siano coinvolti e nel momento in cui abbiano a che fare con l'apparato giudiziario italiano. Lo Stato non riesce più da tempo ad erogare il servizio giustizia in termini che possano definirsi non solo efficienti ma anche solamente accettabili. L'enorme numero dei processi pendenti, l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli con l'incapacità del sistema di gestire anche i soli provvedimenti sopravvenuti stanno determinando e hanno determinato una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia, una sfiducia tale da rendere sempre più concreto il pericolo che si ricorra a forme di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che si incrementi il numero di reati a causa di una sostanziale impunità. Penso che tutti dovremmo essere preoccupati di una situazione di questo tipo, perché Stato di diritto, amministrazione della giustizia e legalità sono i cardini imprescindibili di una convivenza civile, chiunque e qualunque forza politica si trovi a governare il Paese.

Sappiamo tutti che con il cosiddetto processo breve non si possono risolvere i problemi dei milioni di cittadini che chiedono giustizia ogni giorno nelle aule dei tribunali. Questo processo breve instaura un meccanismo a clessidra: finito il tempo, finito il processo; meccanismo introdotto oggi, con queste condizioni date. È per questo che la maggioranza parlamentare si rende responsabile di un fatto gravissimo dando forma e forza di legge ad un permanente diniego di giustizia. Il debito di giustizia che lo Stato ha con milioni di cittadini a causa dei milioni di processi pendenti non solo non verrebbe saldato, ma non sarebbe neppure azzerato: verrebbe reso semplicemente inesigibile, stando ben attenti peraltro a non farlo capire agli elettori, cui si somministra, invece, la solfa falsa che questo provvedimento accelererebbe i tempi. Sono invece milioni i processi che andrebbero a morire, ma si tratterebbe di una morte lenta, di un'agonia strisciante, permanente, incostituzionale e costosissima, perché i processi dovrebbero continuare ad essere celebrati sino allo scadere del termine. Ciò non consente di programmare alcuna riforma. Per questo - ho detto e ripeto - uso l'aggettivo irresponsabile. Il diritto alla ragionevole durata del processo non ha nulla a che vedere con questo processo breve. Il diritto alla ragionevole durata del processo è un diritto di tutte le parti in un processo: è un diritto dell'imputato così come delle persone offese, in nome del quale devono essere portate a termine, a nostro avviso, quelle riforme di sistema, strutturali, costituzionali, ordinamentali e processuali senza le quali la macchina della giustizia non riuscirà a mettersi in moto.

dal caso Tortora in poi e non abbiamo mai cambiato opinione. D'altronde, colleghi, lo stesso ministro Alfano ha dichiarato più volte e cito: «Occorre intervenire sulla giustizia con una riforma organica in tempi rapidi e non con una legislazione alluvionale, ma con interventi mirati che non vanno contro qualcuno sui processi e sull'asse istituzionale‑costituzionale per una giustizia al servizio del cittadino». Queste dichiarazioni però, evidentemente, sono costantemente . Nonostante il Governo abbia accettato una risoluzione proposta alla Camera dalla deputata Rita Bernardini, in realtà abbiamo assistito in questo ultimo anno ad un profluvio di misure che hanno aggiunto fattispecie di reato, che, sull'onda di un imperante populismo demagogico, in realtà convogliano disagio sociale verso i giudici penali e poi verso le carceri, anche loro divenute fuorilegge, illegali e criminogene. Quindi, colleghi, questo provvedimento non ha nulla a che vedere con gli interventi strutturali o con quella grande riforma del sistema giustizia; non ne é neppure l'inizio e anzi, per quanto ne sappiamo, ne é solamente la fine ingloriosa. Aggiungo un'ultima considerazione, che sottopongo all'attenzione di tutti noi, al di là di ipocrisie o di mancanza di coraggio: l'altro elemento che attraversa il sistema sono le oltre 200.000 prescrizioni annuali nel nostro Paese. una forma di amnistia non regolamentata, assolutamente discrezionale e totalmente opaca. C'è da chiedersi se non sarebbe il momento di avere, invece, il coraggio politico d'assumere una responsabilità in Parlamento per un'amnistia che operi sotto l'assunzione di responsabilità e non per prescrizione. Noi tolleriamo un'amnistia e non la governiamo. Mi si dice che ciò avviene perché l'opinione pubblica non lo capirebbe. Questa idea che i cittadini non capiscono

se prima non si dà vita ad una stagione di riforme che permetta alla macchina della giustizia di rimettersi in moto e di entrare a regime con responsabilità e regole nuove, questo processo breve non risolverà la più grande questione politica e sociale del Paese, la più imponente fabbrica di violazioni dei diritti umani e civili, ma sarà capace solamente di risolvere i problemi con la giustizia di alcuni potenti e prepotenti nel nostro Paese, a discapito dei milioni di cittadini che questa sete hanno e questo diritto esigono. *(Applausi dal

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge Gasparri-Quagliariello, comunicato alla Presidenza del Senato il 12 novembre 2009, arriva all'esame dell'Aula esattamente dopo due mesi, già si sono prodotti più emendamenti da parte del relatore, modificandone radicalmente l'impianto in un tormentato *iter*. Il confronto in Commissione giustizia e quello, ancora più ampio, nelle diverse sedi politiche e tecniche, oltre che davanti all'opinione pubblica, hanno dimostrato ampiamente che la stessa maggioranza parlamentare aveva lavorato troppo in fretta sul testo del disegno di legge, pur presentato a suo tempo come intenzionato a risolvere il «problema dei problemi», quello cioè delle interferenze tra sovranità popolare e potere giudiziario, e invece interessato probabilmente solo a liberare il Presidente del Consiglio da uno scomodo appuntamento con la giustizia. Una maggioranza sicura di sé e delle sue ragioni, fino al punto di dichiarare solennemente, per bocca del senatore Quagliariello, «probabilmente saremo costretti a fare da soli», si è poi trovata a dover fare i conti non solo con l'opposizione parlamentare in Senato, ma anche con le critiche di tutte le componenti del mondo giudiziario (Associazione nazionale magistrati, avvocatura, CSM), convergenti nel sottolineare l'incongruità del disegno di legge con le stesse finalità dichiarate. Ragion per cui ci troviamo oggi, all'inizio della discussione generale, sia pur in un tormentato *iter*, a parlare di un testo legislativo che già sappiamo, noi dell'opposizione e voi della maggioranza, che è stato modificato radicalmente. È tuttavia giocoforza, in questa fase, restare al testo in discussione, del quale già nel dibattito in Commissione sono state messe in rilievo le criticità. Non posso però non rilevare che, a quanto risulta dalla semplice lettura dei giornali, la maggioranza non parla più di processo breve, ma preferisce la locuzione «processo certo», che senza dubbio è più aderente al testo dell'articolo 111 della Costituzione, e forse è più accettabile da componenti della stessa compagine governativa meno interessati a difendere, almeno in questo caso, posizioni personali. È stato infatti notato - e mi riferisco al parere sul disegno di legge espresso dal Consiglio superiore della magistratura - che il bene tutelato dalla norma costituzionale, introdotta nel 1999

ma richiede ben altre garanzie per l'imputato e per le stesse ragioni della giustizia. «La fissazione di un termine perentorio per il compimento dei singoli gradi di giudizio che produce l'effetto di estinguere il processo» - ha rilevato nel suo parere il CSM - «non sembra collegarsi alla previsione costituzionale del giusto processo in senso oggettivo, giacché il nuovo strumento privilegia il rispetto della rapidità formale fissata con scansione temporale rigida, non curandosi della necessità che il processo realizzi appieno la funzione cognitiva che lo caratterizza». Alla luce di questa imprescindibile considerazione, la nuova normativa sul processo deve contemperare il diritto di ogni persona a vedere la sua causa esaminata entro un termine ragionevole, ma con il necessario accertamento sul merito della questione dedotta in giudizio. Il diritto consacrato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui il disegno di legge si richiama, e prima ancora dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione, «è anzitutto» - cito ancora il parere del CSM «che il processo ci sia e che sia un processo che si concluda con una decisione di merito. In secondo luogo, che sia un processo di durata non irragionevole ed improntato agli altri principi descritti dalla norma costituzionale». A questi criteri ci si deve attenere nel valutare il presente disegno di legge. E in base a questi criteri non si può non rilevare che il testo che stiamo esaminando definisce, sì, i tempi di durata dei diversi gradi di giudizio, ma non garantisce, né potrebbe farlo, che alla scadenza prefissata si pervenga ad una decisione di merito. C'è un'evidente contraddizione tra un'astratta predefinizione dei tempi e la certezza di arrivare a sentenza, ed è proprio per questo motivo che si è giustamente parlato di questa legge come di un provvedimento di "amnistia generalizzata" che il Parlamento approverebbe come legge ordinaria, senza la prescritta maggioranza qualificata. Ciò vale, è bene dirlo da subito, anche nel caso in cui la maggioranza parlamentare, facendo proprie una parte delle critiche di cui il disegno di legge è stato fatto oggetto, mutasse alcuni termini della questione eliminando con appositi emendamenti, come è avvenuto e come si appresta a fare, le parti più macroscopicamente irrazionali del testo, che sono l'esclusione di alcuni reati - e dei più gravi - o di alcuni imputati - i recidivi - dal computo di tempi del cosiddetto processo breve, o modulando diversamente i tempi entro i quali devono obbligatoriamente svolgersi i gradi di giudizio. Il problema non è questo: il problema è che perché il processo sia "giusto" e anche ragionevolmente "breve", occorre garantire alla macchina giudiziaria le condizioni perché sia possibile giungere all'accertamento processuale dei reati. Tutto ciò non è previsto dal disegno di legge in esame, che infatti non si cura assolutamente di focalizzare il vero tema della riforma della giustizia affrontando materie quali gli organici della magistratura e degli uffici giudiziari, la riorganizzazione delle circoscrizioni, la depenalizzazione dei reati minori, il ricorso alla conciliazione: interventi e riforme che potrebbero garantire, se attuate, un processo breve e giusto. Ma, mi chiedo, i tempi diversamente i tempi diversamente distribuiti consentiranno di arrivare a sentenza? E se non si arriva a sentenza, è giusta la prescrizione dei processi, l'annullamento dei diritti? La prescrizione dei processi è moralmente accettabile? È sostenibile, dal punto di vista della moralità pubblica, una prescrizione che non dà una risposta alla domanda sul diritto leso, compromesso, negato? Dietro il processo "breve" o "certo", comunque la maggioranza voglia definirlo, si nascondono problemi personali ben individuabili. Ho l'impressione che si voglia arrivare ad un'amnistia mascherata e che non si abbia il coraggio di assumere una posizione netta. Chiedo al Governo: si vogliono garantire i vertici, o solo uno di essi, degli organi costituzionali? Bene, allora si faccia una norma costituzionale. Contingentando i tempi, in una democrazia che funziona, per approvare una norma costituzionale, con doppia lettura di Camera e Senato, basterebbero cinque mesi. Se invece si vuole un "lodo", al riparo dalla decisione della Corte costituzionale, la maggioranza abbia il coraggio di chiederlo al Parlamento, senza ipocrisie e sotterfugi dannosi per il Paese e la nostra democrazia.

Per la verità, quando è stato presentato questo disegno di legge e ne ho letto il titolo: letto il titolo: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione

Si aspetta che lo Stato abbia l'intenzione, finalmente, di migliorare un servizio essenziale che deve rendere ai propri cittadini: il servizio giustizia. Lo dico a che sostiene che non è indispensabile che un processo cui si dà inizio si concluda con una sentenza che, in sede civile, dica chi ha ragione e chi ha torto e, in sede penale, se un cittadino che è stato accusato di un reato è innocente o colpevole. Non si deve dire più questo,

da una giustizia lenta, che arriva in tempi inadeguati, ad una denegata giustizia. ad una denegata giustizia, perché, quando si estingue il processo, si nega la giustizia al cittadino, che si è rivolto allo Stato per sapere se ha ragione o torto in una causa civile.

E allora è lo Stato che rinuncia a dare giustizia ai cittadini. Ricordo di aver letto nei libri, quando ero all'università, che il servizio si dava ai cittadini *ne* *cives* *ad* *arma* *ruant*. Era questa l'espressione che si usava, perché, quando lo Stato non dà giustizia ai cittadini, questi ultimi si fanno giustizia da soli, con le armi, se necessario.

Quando lo Stato non è in condizione di rendere giustizia, la gente si rivolge alla criminalità organizzata: è questo il grande cancro che affligge il Sud dell'Italia.

ed esercitava a Napoli, occupandosi prevalentemente di cause di sfratto; ad un certo punto ha dovuto cambiare quasi completamente la sua attività, perché subentrò la camorra. Era molto più facile andare dalla camorra, per ottenere la casa che spettava per urgente ed improrogabile necessità. La camorra andava giù prendeva chi non se ne voleva andare: la prima volta lo avvertiva e la seconda volta lo riempiva di botte. Il terzo giorno, questa persona se ne andava tranquillamente. Vogliamo fare questo? Vogliamo ridurre l'Italia in questo stato? Da quello che ho letto, dalla relazione redatta dagli studiosi del processo

ci siamo lamentati di questo), è stata esercitata l'azione disciplinare e gli impiegati corrotti non sono stati cacciati dall'amministrazione, per questa ragione. È una cosa diversa, che riguarda la dignità delle persone che appartengono ad una determinata amministrazione. Lo sappiamo, lo abbiamo visto anche nel l'unica amministrazione che cacciò i piduisti fu la magistratura. Li hanno fatti condannare tutti e li hanno espulsi dalla magistratura. chi è stato condannato e chi invece se ne è andato per conto suo, perché ha saputo che non si voleva questa gente nella magistratura. Ci stiamo comportando Ci stiamo comportando come se non sapessimo quali sono le ragioni per cui i processi in Italia durano per un tempo intollerabile. Abbiamo 5 milioni di processi civili e 5 milioni di sopravvenienze. Abbiamo la più alta litigiosità. Abbiamo - come si è visto - 3.800.000 processi penali, con i magistrati distribuiti sul territorio in una maniera folle,

tra il processo accusatorio, con la giuria e con l'esecutività della sentenza di primo grado, e un processo che non è accusatorio, ma che non è «né carne né pesce». Abbiamo stabilito che la prova va raccolta in dibattimento e abbiamo inserito questa disposizione anche in Costituzione, all'articolo 111: abbiamo quindi spostato tutto sul dibattimento. Abbiamo fatto affidamento, per questo, sui riti alternativi, che non hanno funzionato. Lo sappiamo tutti, tant'è vero che oggi, da più parti, si chiede anche l'abolizione del rito abbreviato, proprio perché con tale rito non si può più neanche combattere la criminalità organizzata,

perché ci rendemmo conto che non si poteva svolgere un'udienza preliminare trasformandola in una specie di giudizio di primo grado secondo il

abbiamo trasformato l'udienza preliminare - che doveva essere un'udienza filtro per andare subito al dibattimento davanti al giudice naturale, in cui raccogliere la prova - in un'udienza secondo il

e rinvia. Signori, siamo qui in un'Aula vuota: evidentemente la giustizia a questo Paese e a questa maggioranza non interessa più,

erroneamente. A questo punto non siamo più in un Parlamento, ma in un ammasso. Allora, signori cari, se vogliamo continuare continuare senza tener conto neanche di questo, ricordate che a quelle prescrizioni che vi sono state indicate dal Ministro si aggiungeranno queste forme di prescrizioni. L'altra questione di legittimità costituzionale che desideravo muovere al

Premesso che, per evidenti ragioni, parte delle riflessioni che andrò a sviluppare riguarderà anche il contenuto degli emendamenti presentati dal relatore, che costituiscono una preziosa traccia che chi sta parlando integralmente condivide, vorrei intanto rassicurare il collega D'Ambrosio su due aspetti fondanti. Il primo è che chi sta parlando in questo momento, e che con grande attenzione lo ha ascoltato, è abituato a ragionare da sempre con la propria testa, così come tutti coloro che siedono su questi banchi. Infatti, se la logica dovesse essere quella delle lucine che si accendono, ahimè, quanto detto dal senatore D'Ambrosio sarebbe ampiamente reversibile e rovesciabile su chi siede sui banchi dell'opposizione, perché parimenti ciò regolarmente accade. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che questa maggioranza ha particolare riguardo ed attenzione ai problemi della giustizia, proprio perché vuole evitarne un uso strumentale che sin troppo bene conosciamo.

che il cittadino, per quanto possibile, non debba più pagare i costi personali, e non solo personali, del disservizio della giustizia. In secondo luogo, con grande franchezza e onestà intellettuale, mi chiedo quanta parte vi sarebbe dell'apparente tensione ideale che caratterizza questo dibattito e dell'acrimonia che in qualche misura ne ha contraddistinto alcune fasi, e solo di merito si andrebbe a parlare, laddove queste norme non potessero anche riguardare vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio, che è un cittadino della Repubblica italiana come tutti, cosa che non va mai dimenticata. Dico questo perché ciò che noi stiamo facendo è il primo concreto tentativo di dare attuazione ad un precetto costituzionale: la ragionevole durata del processo. Nessuno parla in termini di processo breve; anzi, se dovessi riprendere le parole del collega Li Gotti, certamente non breve potrebbe definirsi quel sistema che faticosamente, faticosamente, soprattutto grazie anche all'attenta rilettura che il relatore ha fatto di tutto ciò che è scaturito nel dibattito in Commissione e all'esterno di questo Palazzo. precetto che fino ad oggi, piaccia o no, è rimasto totalmente inattuato. Questa è la prima grande carenza con la quale ci dobbiamo necessariamente confrontare e coraggiosamente ci stiamo confrontando. L'altra, che è una situazione assolutamente emergenziale e che comunque certamente non giova alla dignità e all'immagine del Paese, è l'innumerevole serie di pronunce della Corte europea di condanna nei confronti del nostro Paese, proprio in relazione a questo aspetto del quale stiamo parlando e ai costi spaventosi della legge Pinto, che comunque necessariamente non possono essere misconosciuti e trascurati, né ulteriormente aggravati. Che sia stato e sia un problema di cogente risoluzione è stato opportunamente e ripetutamente ricordato in quest'Aula. Bene ha fatto il collega Mazzatorta a leggere alcuni passi riconducibili ad una delle più autorevoli figure che hanno contraddistinto la presenza del centrosinistra in quest'Aula; un autentico galantuomo del diritto, come possiamo definire Elio Fassone, già anni fa aveva teorizzato la necessità, proprio in virtù anche della peculiarità della situazione giudiziaria italiana, di individuare un istituto che in qualche modo a quel precetto costituzionale desse una sua oggettiva attuazione. C'è stato un *iter* particolare per quanto riguarda questo disegno di legge. In una prima fase, che potremmo definire più prudenziale, si è

fermo restando, un aspetto che non è superabile se non vogliamo parlare in termini generici, trasformando il nostro dibattito e ciò che andremo eventualmente a produrre sul piano normativo in una grida manzoniana inattuabile. Mi riferisco al fatto che i criteri non possono che essere oggettivi, perché altrimenti, al di fuori di un'oggettivizzazione dei criteri, la ragionevole durata del processo rimane un bel principio destinato ad essere costantemente inattuato, perché delegato ad una mera valutazione potestativa caso per caso.

Questo opportunamente ha fatto il relatore, nell'applicazione di un criterio che è *erga omnes*, ma modulato con varie fasce e con tempistiche diverse, tenendo anche conto del fatto

su basi paritarie è ugualmente dettato costituzionale ancora inattuato in questo Paese e si è fatto di tutto perché le parti non fossero in posizioni di parità: su questo la magistratura - lo ripeto - ha responsabilità gravissime, che non possono essere sottaciute.

Quindi non è neppure vero che vi sia una denegata giustizia da questo punto di vista e che il processo non possa concludersi con sentenza: è vero esattamente il contrario, posto che l'imputato intenda comunque essere definitivamente processato fino alla conclusione del processo stesso.

non è provvedimento riconducibile all'attuale maggioranza - sarebbero stati comunque destinati al macero e ad ingolfare ulteriormente una macchina della giustizia che già arranca penosamente, schiacciata tra l'altro proprio dal peso di quanto abbiamo detto.

non sono i collaboratori di giustizia che parlano ad orologeria ma è questo Governo che opera ad orologeria: questo provvedimento non è certo tra i *desiderata* degli italiani. Crisi, disoccupazione, formazione, casa, sviluppo ridotto, imprese al tracollo, scuola, criminalità organizzata e prospettive per le nuove generazioni provocano l'insonnia dei nostri connazionali. Invece voi, maggioranza e Governo, dovete spiegare le ragioni di un provvedimento che manderebbe in prescrizione reati gravissimi. Ma per voi sono bazzecole. Distruggete il sistema giudiziario con la più grande amnistia, collega Mugnai, una scelta irragionevole, un provvedimento che vìola i principi di uguaglianza di fronte alla legge perché si applica anche a reati gravissimi. Qual è l'urgenza per il Paese? È a rischio la vita o l'incolumità di un ragguardevole numero di italiani? Certo che no. Ha ragione la presidente Finocchiaro quando si chiede quanti innocenti non vedranno dichiarata la loro innocenza a seguito di un processo regolare e quanti colpevoli non verranno assicurati alle patrie galere in relazione a delitti comuni. Ma ciò che è più tragico, e che potrà accadere con un semplice calcolo degli eventi, è che si introdurrebbe un incentivo a violare la legge sapendo di poter contare su un'alta probabilità di farla in barba alla legge stessa, soprattutto nelle grandi città. A Palermo, nel tribunale, in una della procure più impegnate nella lotta alla criminalità mafiosa, a fornire una spiegazione possono concorrere alcuni dati sul sistema giudiziario e sul personale In corte d'appello su 66 magistrati ne operano solo 47; degli 88 giudici di pace ne mancano all'appello 28; nella magistratura ordinaria non togata la scopertura è del 32 per cento; nell'organico del personale amministrativo su 1.830 dipendenti previsti ne mancano 293; 55 dovrebbero essere i direttori di cancelleria ma solo 38 operano; 17 i cancellieri sui 72 previsti. Ma con il processo breve quanti mafiosi verranno liberati? Un collegamento audio‑video saltato, un trasferimento ritardato da un penitenziario al tribunale... Insomma, un provvedimento senza risorse adeguate: si darebbe quindi la stura a quella che chiamo la mega-amnistia. Con questo provvedimento si vogliono sovvertire le regole della ragionevolezza e tutto ciò si inserisce in un disegno ampio di stravolgimento della Costituzione. È plausibile pensare che si voglia creare una classe di persone che sapranno di poter confidare su un sistema che consentirà loro di perseguire il proprio interesse contro la società. Si crea di fatto un *vulnus* che aumenterà il dubbio tra il rispetto della legge e la perpetrazione del reato, visto che chi delinque in molti casi non pagherà nessun prezzo. Volete il processo breve *ad personam*, ma è la Costituzione che esige che il processo abbia una ragionevole durata. Ecco perché è necessario che la riforma dei tempi si valuti tenendo conto della ricaduta sulla generalità dei processi. Ma c'è una volontà sovrana del popolo che è la condizione necessaria per sottrarre, secondo voi, ma anche e soprattutto secondo lui, il *Premier* alla comune uguaglianza giuridica che lega tutti i cittadini di una Nazione democratica. Ma il *primus super pares* vive un'eccezionalità ed una straordinarietà che gli sono dovute dal suo *status*. L'eletto, il divino, è oltre l'ordinamento giuridico. Anziché condividere una norma generale che intervenga sulla durata irragionevole del processo, si mettono i piedi nel piatto. Con questo provvedimento, un incensurato che mette in campo una truffa milionaria può farla franca se il processo non si conclude in due anni, mentre per un recidivo, morto di fame, che commette una truffa per pochi euro il processo non finisce mai fino a che non arriva la condanna. Ma ormai avete scelto, avete obbedito al *diktat* degli onorevoli avvocati del Premier. È un momento nero per la giustizia italiana e anche per chi combatte la criminalità organizzata la mafia. Ci troviamo di fronte ad un combinato disposto che rischia di far arretrare anni di conquiste dello Stato e della società e contestuali sconfitte per il crimine organizzato. Avete nelle mani una bella scala reale che cedete che cedete alle organizzazioni criminali: processo breve, intercettazioni, scudo fiscale, vendita dei beni confiscati, azzeramento fondi per le parti civili, le associazioni e gli enti pubblici che affiancano le vittime di mafia. Riducendo le intercettazioni per alcuni reati ne riducete il rango di prova annullandone il valore probatorio. Con lo scudo fiscale, con molta probabilità, altre mafie investiranno in immobili nel nostro territorio, magari in quelli confiscati alla mafia. Vi fregiate degli arresti dovuti grazie a magistrati, carabinieri e polizia e poi non pagate gli straordinari alle forze dell'ordine. La sezione catturandi di Palermo si è autotassata per far fronte alle spese necessarie per arrestare il numero due di Cosa Nostra. Mettete i beni confiscati all'asta per fare cassa. Ma chi parteciperà all'asta se non i mafiosi e i loro prestanome? Leggete le novelle rusticane di Verga del 1858. Mazzarò difende la "roba", che per lui è ricchezza, potere ma anche simbologia di forza, come per i mafiosi.

intervengo sul provvedimento senza dimenticare le povere popolazioni di Haiti che sono state sterminate dal terremoto.

cittadini. Sappiamo quanto risulti complicato e addirittura tormentoso tentare di porre mano alle necessità della giustizia in Italia. difficoltà che ritroviamo in questa circostanza, alimentate o scaturite dal fardello di soggettive valutazioni circa le motivazioni che avrebbero spinto a legiferare in materia di ragionevole durata dei processi. Stentiamo ad abbandonare il campo delle dietrologie quando, con maggiore oggettività, potremmo innanzitutto attenerci al titolo del disegno di legge in discussione, il quale colloca questo provvedimento nell'ambito degli atti dovuti. Il titolo, infatti, recita: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Si tratta, dunque, di ottemperare ad obblighi precisi, tesi a garantire il funzionamento della giustizia. Non è forse questo lo spirito che indusse, nel 2004 come nel 2006, gli allora DS a presentare una proposta di legge per introdurre quello che, nell'attuale circostanza, chiamiamo processo breve?

ritengo che, nella coscienza *bipartisan* di una esigenza tanto diffusa, la prospettata riforma si debba valutare per le ricadute che comporterà nell'esistenza di milioni di persone, piuttosto che per gli effetti eventualmente prodotti nell'ambito di qualche contenzioso eccellente. Eppure dai *media* apprendo di perplessità dei parlamentari, magari anche della maggioranza, nel sostenere questo provvedimento, bollato come garantista proprio perché letto e interpretato alla luce di note e controverse vicende giudiziarie. Ma è garantismo far si che il cittadino accusato di un reato ottenga la sentenza definitiva nello spazio di sei anni? È garantismo permettere che le vittime dei reati non attendano all'infinito l'ora della giustizia? E soprattutto è garantismo chiudere il mortificante capitolo delle lentezze e negligenze giudiziarie, autentica fabbrica di impunità e iniquità? Sappiamo che i delitti di mafia, insieme ad altre fattispecie dette di particolare allarme sociale, sono stati compresi nel provvedimento con una durata più lunga. I signori magistrati potranno continuare a lavorare su queste vicende con la ponderatezza usuale; per lo scalpore che suscitavano, furono precisamente le lentezze e le distrazioni compiute dagli addetti ai lavori nei procedimenti antimafia a rompere il silenzio sulle inefficienze della nostra giustizia nel suo complesso. Tra i tanti analoghi penso ad un episodio dell'aprile dell'anno scorso, senatore D'Ambrosio, e alla GIP barese che già da un anno avrebbe dovuto depositare le motivazioni della sentenza relativa alla condanna di 21 presunti boss mafiosi. Nonostante il ritardo, chiede una proroga di 90 giorni che le viene concessa; trascorsi i tre mesi ne chiede un'altra, concessa anche questa; quasi al termine del periodo utile le giunge la promozione a presidente del tribunale dei minori. Lascia l'incartamento al collega che le subentra, il quale domanda subito una proroga di 90 giorni che, naturalmente, gli viene accordata. Da una proroga all'altra, alla fine, scadono i 15 mesi della carcerazione preventiva e i 21 presunti boss mafiosi possono tornare in libertà. Grande scandalo, grancassa mediatica, altisonanti proclami, ma nei confronti della GIP non scatta nessuna sanzione. Come al solito si incolpano le carenze della struttura, visto che, secondo il CSM, in quella sede mancava chi avrebbe dovuto ricordare al magistrato la scadenza del proprio lavoro. Tutto questo è accaduto in un tribunale ad elevata informatizzazione. Capite bene, colleghi senatori, come diventi arduo coniugare questa riforma all'equazione più fondi uguale prestazioni migliori, che pure è stata riproposta nell'attuale circostanza. Cifre ben conosciute attestano che per risorse destinate alla giustizia lo Stato italiano non si discosta dagli altri Paesi europei, ma nel bel Paese questi fondi vengono assorbiti più che altrove dalla voce stipendi dei magistrati Nel momento in cui si pretendono sacrifici dai cittadini e miracoli di produttività da tanti malpagati lavoratori, credo si possano sollecitare dai giudici risultati diversi da quelli che ci hanno sprofondato ai posti più bassi nelle classifiche internazionali dell'efficienza giudiziaria. Dei 47 Stati che compongono il Consiglio d'Europa, solo Bosnia e Croazia evidenziano una giustizia più lenta. Lo stesso organismo comunitario, periodicamente, pubblica il rapporto sulla qualità della giustizia dei Paesi europei, offrendo impietosi raffronti. Cito a titolo di esempio i nostri 3.688.000 processi civili pendenti contro il milione di cause pendenti in Francia, nazione con numero di abitanti pari al nostro, mentre in Germania non si raggiunge il mezzo milione. Tali classifiche, apparentemente virtuali e simboliche, trovano concreta rispondenza nella vagonata di milioni che lo Stato regolarmente sborsa quali penalità e indennizzi per i danni causati alle persone e alle imprese dagli inammissibili ritardi della giustizia. In questo senso, a chi paventava la cancellazione di 100.000 processi per effetto del provvedimento in oggetto si sarebbe potuto contrapporre altrettanto sgomento per la supposta esistenza di questi 100.000 procedimenti che la magistratura italiana non riesce a chiudere in sei anni. Tuttavia, e concludo, poiché non smetteremo mai di credere nel valore assoluto della giustizia, prendiamo atto con soddisfazione di come le ultimissime modifiche apportate al disegno di legge, oltre a superare qualche obiezione di incostituzionalità, riducano ragionevolmente l'ambito dei processi a rischio di estinzione per effetto della nuova normativa. Tale soluzione è anche frutto di un confronto politico che il nostro movimento non si stanca di sollecitare, nella consapevolezza che riforme vere e destinate a incidere nella vita delle persone non possano prescindere dal più ampio coinvolgimento di quanti, al di là degli schieramenti, sono chiamati ad operare per il bene dei cittadini.

onorevoli senatori, finalmente possiamo parlare di processo breve in un'Aula di Parlamento. Fino a ieri abbiamo ascoltato l'annuncio che ne è stato fatto sulla stampa solo pochi mesi fa, dopo che la Corte costituzionale

Abbiamo seguito i commenti della stampa internazionale e ci siamo attentamente interrogati, con la dottrina dei migliori giuristi del nostro Paese, sulla fattibilità e sull'utilità concreta delle norme per accelerare lo svolgimento del processo penale che giustamente, si è detto, in Italia supera di molto tempi ragionevoli. Praticamente abbiamo trascorso tutto questo tempo - non tanto, poi, se si pensa alla pronta fissazione nel calendario d'Aula

Ora interveniamo su un testo sapendo, come spesso accade con questo Governo, che il testo esaminato in Commissione e portato poi alla discussione dell'Aula ha subito profonde modifiche e non a seguito dell'attività emendativa parlamentare, ma è stato corretto, limitato e valutato a prescindere dal dibattito parlamentare, solo per la sua capacità di produrre l'effetto principale per cui è stato pensato e cioè salvare l'imprenditore Berlusconi, ora Premier del nostro Paese: salvarlo dal processo Mills e da quei processi che, a vario titolo, ha accumulato nel corso della sua vita imprenditoriale. comunque, obbligata a seguire questo percorso irrituale in Parlamento, mi sono ripromessa di intervenire affrontando non tanto il tema sul piano giuridico-legislativo, ma cercando invece di valutare l'impatto sociale e politico di queste norme nel pianeta giustizia, nel sistema Paese. Propongo tre punti alla riflessione dell'Assemblea. Per Per semplificare al massimo il concetto parto con una domanda. Senatore Valentino, quanto dura un processo in appello? Quanto tempo prende la trattazione in aula di un processo nel secondo grado? Chi è pratico di aule di giustizia sa che, salvo rare eccezioni, un processo dura in media da mezz'ora a due ore, a seconda dei tempi che utilizzano la procura generale o i difensori per spiegare le loro ragioni giuridiche. Credo che possiamo dire che nel 90 per cento dei casi la fase dell'esame pubblico, dibattimentale dell'appello non supera le due ore di tempo. Questo vuole dire che il tempo che va da quelle poche ore ai tempi previsti da questo disegno di legge è utilizzato per le notifiche, per la stesura della sentenza e soprattutto dal carico dei processi, cioè dalla quantità dei processi da trattare e dalla burocrazia a difesa delle garanzie. Insomma, ho fatto un conto tenendo in considerazione le norme processuali vigenti. Seguendo le norme attuali si potrebbe celebrare un processo d'appello in quattro mesi, tenendo conto dei soli tempi processuali. Di questi quattro mesi per il processo vero e proprio, come abbiamo detto, servono nella media due ore (mi sono tenuta molto larga). Quindi, i due o tre anni attuali sono imputabili all'insufficienza dei mezzi messi a disposizione del sistema giustizia. Possiamo dunque affermare che, se la macchina avesse i mezzi per lavorare di più (cancellieri, cancelleria, carta per le fotocopie, giudici che fanno udienza tutti i giorni per tutto il giorno), i tempi della giustizia italiana verrebbero drasticamente abbattuti. Ho fatto l'esempio del grado di appello, ma, *mutatis mutandis*, potrei farlo per la Cassazione. Diverso è invece il primo grado, che richiede tempi e riti diversi a seconda della complessità della materia trattata e del numero degli imputati o testi necessari alle parti. Credo fermamente, però, che anche in primo grado una migliore efficienza del sistema possa abbattere drasticamente i tempi processuali. La conclusione politica sull'esempio processuale porta direttamente alla responsabilità di questo Parlamento: il problema non è fissare un tetto temporale ai processi superato il quale questi ultimi si prescrivono, ma è quello di creare le condizioni perché essi si possano svolgere nel più breve tempo possibile. Questo è compito del Parlamento e non dei giudici. I giudici applicano le leggi, ma è il Parlamento che decide quali leggi. A conferma di quanto ho detto si può leggere oggi, sulla prima pagina del «Corriere della Sera», il caso di Cassano d'Adda, dove la mancanza di un cancelliere

senza altre valutazioni sulla pericolosità, sulla gravità dei fatti e sull'impatto che produrrà, soprattutto in alcune zone del Paese. Sappiamo che per evitare problemi di costituzionalità le norme sono state estese anche ai recidivi.

Siamo invece interessati a compartecipare alla discussione ed alla votazione di qualsiasi norma migliorativa dell'attuale assetto. Credo che, dopo tutti i tentativi che avete messo in cantiere per introdurre norme «salva Berlusconi imprenditore», utilizzando le norme generali di un codice che aveva riconosciuto a livello internazionale una tradizione giuridica motivo di vanto per il nostro Paese, sia ora di fermarvi e riconoscere pubblicamente che avete un problema da risolvere:

Ma non modificate un sistema (che peraltro va modificato) con norme che, anziché agevolare lo svolgimento dei processi, mettono un cartello con scritto «peccato, fine della corsa».

vorrei occuparmi della questione principale, ossia degli effetti che la normativa in esame dovrà produrre sul sistema giudiziario.

nei presentatori del disegno di legge, nonché nei componenti e colleghi della maggioranza,

portare con sé l'aspirazione e anche il convincimento che molti sono gli effetti che la legge produce. Invece c'è un tentativo per essere rassicurati lungo questa strada. Ora, se non ne dovesse produrre tanti e quindi dovessimo riscontrare come ragionevolmente fondata l'opinione della maggioranza, dovremmo dire che siamo in presenza di una norma inutile; oppure, come nel caso e nella valutazione che noi ne facciamo, che siamo in presenza di una norma preoccupante, perché non risolve nessuno dei problemi della giustizia. Non li risolve, come

dettame normativo che si occupa di sottrarre giustizia e non di offrirne a coloro che la rivendicano.

Signor Presidente, le opposizioni ritengono che la causa di tutti i mali della giustizia italiana sia riferibile alle politiche del Governo di centrodestra. Voglio ricordare agli immemori che il centrosinistra ha governato il nostro Paese nella legislatura dal 1996 al 2001 e in quella dal 2006 al 2008, se oggi il centrosinistra non è al Governo è perché è stato rimandato a casa dagli elettori. È proprio questo il problema. Da parte delle sinistre si cerca per via giudiziaria di stravolgere il risultato elettorale del 2008. Dobbiamo dire le cose come stanno. Quando il senatore D'Ambrosio individua tra le cause o, quantomeno, come causa principale dei guasti della giustizia italiana il codice di rito del 1989 dimentica però di aggiungere che di quel codice noi non siamo assolutamente responsabili. Non c'era nel 1989 Alleanza Nazionale, non c'era Forza Italia e men che mai c'era il Popolo della Libertà. C'era il Movimento Sociale Italiano relegato all'opposizione, però c'era il Partito Comunista Italiano, prima, e il Partito Democratico della Sinistra, poi, che storicamente sono i vostri partiti di riferimento. che vi sia una crisi della giustizia l'ha riconosciuto anche lei, senatore D'Ambrosio, e non poteva non farlo. I processi pendenti nel nostro Paese sono quasi 9 milioni:

Sono dati ufficiali noti a tutti noi. Il confronto con i nostri vicini europei è davvero impietoso. Nel 2006 non lo dico per malizia, sapendo che nel 2006 voi eravate al Governo, lo dico perché è un dato statistico di cui sono in possesso, in quanto fornito dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia - le cause civili pendenti

La situazione peggiora se consideriamo le cause pendenti in tribunale in sede penale. Qui da noi, sempre nel 2006, quando voi eravate al Governo, erano 1.200.000; circa cinque volte in più rispetto alla Germania, quindici volte in più rispetto al Regno Unito. Come ha ricordato il professor Vincenzo Carbone, primo presidente della Suprema corte di cassazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel gennaio dell'anno scorso, in media occorrono poco meno di mille giorni (960 per la precisione) per ottenere giustizia nel nostro Paese: tre anni per poter avere un giudizio in primo grado nel civile, 1.509 giorni per un giudizio in appello, 426 giorni per un giudizio di primo grado nel penale, 730 per un giudizio di appello. Potrei continuare ancora; ma questi sono dati assolutamente incontestabili. Questa crisi evidentissima ci ha cagionato - come ha ricordato giustamente il senatore Mugnai - ricorrenti condanne dalla Corte europea per i diritti dell'uomo.

nel penale, centinaia di migliaia di processi che vengono travolti dalla prescrizione del reato. Questo Governo, in poco più di un anno e mezzo, ha fatto quello che voi non avevate mai fatto. Abbiamo realizzato e completato la riforma del processo civile. Dopo decine e decine di anni,

introdotto nel nostro ordinamento le misure più severe nei confronti della criminalità organizzata, colpendone i patrimoni, cosa che mai in precedenza si era verificata. infine, in Commissione giustizia del Senato, la grande riforma del processo penale. Noi non abbiamo mai sostenuto - non l'ha fatto il senatore Valentino, non l'ho fatto io e non l'ha fatto nessuno di questa maggioranza di questa maggioranza - che il disegno di legge attualmente al nostro esame rappresenti la grande riforma della giustizia italiana. Esso è un tassello di una riforma molto importante, che noi dobbiamo approvare come Parlamento e che approveremo di sicuro, perché è nel programma del Popolo della Libertà. a sua volta, fa parte di una grande riforma, che deve aggiungersi come riforma istituzionale, come riforma del fisco e come riforma in termini di sicurezza. Colleghi, opposizioni avete aprioristicamente criticato il centrodestra per questo disegno di legge, che inizialmente prevedeva due anni per il primo grado, due anni per l'appello e due per la Cassazione.

(il senatore Maritati, attuale senatore e vice presidente della Commissione giustizia, fu uno dei firmatari) - proponeste una legge sostanzialmente analoga a quella che era stata presentata: due anni per il primo grado, due anni per l'appello, due anni per la Cassazione. Potreste dire che nel 2001 vi siete sbagliati; ma nel 2006, quando voi eravate al Governo, un altro gruppo di autorevoli senatori dei Democratici di Sinistra, tra cui l'attuale presidente del Gruppo del Partito Democratico, la senatrice Anna Finocchiaro, ripresentarono il medesimo disegno di legge, secondo lo schema "due anni più due anni più due anni", perché vi eravate resi conto

tutti: voi vorreste una riforma valida per tutti i cittadini italiani tranne che per Silvio Berlusconi. Questa è la verità. Voi ci accusate di approvare delle norme *ad personam*, voi vorreste una norma *contra personam*, valida per tutti i cittadini italiani eccetto uno: Silvio Berlusconi. Se questa è democrazia, è una democrazia che lasciamo volentieri a voi. Il senatore Valentino ha presentato una serie di emendamenti che certissimamente migliorano l'impianto del disegno di legge arrivato in Commissione giustizia, raccogliendo le obiezioni più serie che erano state sollevate sia dalle opposizioni che all'interno della stessa maggioranza. Perché, vedete, quell'impianto lasciava delle forti perplessità in termini di compatibilità costituzionale. Quei dubbi, che noi avevamo e che voi avevate, sono stati risolti brillantemente dal senatore Valentino, che ha eliminato qualsiasi impropria distinzione tra imputati incensurati e imputati censurati, perché quando si va a colpire il procedimento, è chiaramente non apprezzabile il fatto che si faccia una distinzione tra imputati. Nello stesso tempo, c'erano dei reati inseriti impropriamente, in una sorta di fiera delle occasioni: giustamente il senatore Valentino li ha tolti di mezzo. Si dice - è stato detto anche oggi pomeriggio - che il disegno di legge, se venisse approvato, determinerebbe dei guasti incredibili e non quantificabili. realtà è meglio non parlare, caro senatore Valentino, di processo breve, perché il processo che è al nostro esame tutto si può definire tranne che processo breve. Quando pensiamo che un giudizio per un reato con pena edittale massima inferiore a dieci anni deve durare tre anni in primo grado, due anni in appello, un anno e mezzo in Cassazione e, in caso di annullamento con rinvio, un anno per ogni ulteriore grado di giudizio e arriviamo ad una durata di nove anni e mezzo, senza considerare il tempo occorrente per le indagini preliminari; se prendiamo l'ipotesi di un reato con pena edittale pari o superiore a dieci anni, i nove anni e mezzo diventano dieci anni e mezzo; se prendiamo i reati più gravi,

per reati indultabili in base alla legge del 2006? Si tratta di quei reati per i quali, come giustamente ha ricordato il senatore Valentino questa mattina in Commissione giustizia, mai e poi mai il condannato andrebbe a scontare la pena: tra i tre anni di indulto e gli altri tre anni di affidamento in prova ai servizi sociali in base all'ordinamento penitenziario, va da sé che nessun cittadino italiano andrebbe in galera per un reato indultabile. Voglio ricordare, infine, che il procuratore Maddalena, con la sua famosa circolare, diede indicazioni comportamentali ai procuratori della Repubblica. La circolare Maddalena, del 10 gennaio 2007,

pur nell'eventuale epilogo di una sentenza di condanna, avrebbero visto la pena inflitta non concretamente applicata o applicabile; quindi, il procuratore Maddalena

cento degli italiani è interessato alle riforme costituzionali, poco più del 20 per cento è interessato ai problemi legati al lavoro

intervengo per parlare ancora una volta in quest'Aula del problema legato alla FIAT di Termini Imerese. hanno scioperato, recandosi davanti al palazzo della Presidenza dell'Assemblea regionale e poi all'Assemblea regionale stessa. Sono dell'avviso che le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato Marchionne abbiano creato un momento di

indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», introduce nell'ordinamento